link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Dopo l'audizione delle parti sociali e la discussione in Commissione, la relatrice ha fatto una buona sintesi della volontà espressa, cercando un massimo comun denominatore tra le parti ed inserendo correttivi al provvedimento rispetto a quanto arrivato dalla Camera, che sicuramente chiariscono ed implementano il provvedimento stesso. L'Italia dei valori, che di legalità e giustizia ha fatto un *mantra*, crede che questo provvedimento sia un passo ulteriore, seppur timido, verso la giustizia sociale. Sicuramente poteva essere migliorato, ad esempio attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, tra i quali quello della senatrice Bignami, che verteva sull'8 per mille da destinare al fondo che viene istituito In tutti i casi, credo che quello che non siamo riusciti ad inserire oggi possa comunque essere preso in considerazione dal Governo, magari nella prossima legge di stabilità. Oggi l'8 per mille è dedicato a tipologie di interventi quali la fame nel mondo, le calamità naturali, la conservazione dei beni culturali e l'edilizia scolastica con delibera del Consiglio dei Ministri, è stata prevista l'assegnazione di una quota parte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare, in questa fase di emergenza, l'operatività dei centri di accoglienza. Quindi è stato aggiunto un ulteriore capitolo. Spero che in futuro una quota parte di questo 8 per mille possa essere dedicato a fondi *welfare*, quali quello per la disabilità grave o quello per le vittime di reati di violenza intenzionale.

Presidente, signori senatori, voterò «no» al *referendum* della vostra "schiforma" costituzionale.

ha migliorato e ne ha cambiato, anche se di poco, la sostanza. Innanzitutto devo distinguere il merito dei principi e il merito dei fondi. Dopo le dichiarazioni dei giornali di oggi, dove sembra che il ministro Padoan si accinga a chiedere un altro aiutino all'Europa, credo sia meglio acchiappare Per il merito dei principi, invece, ho sempre l'idea che sarebbe bastato mettere 100 milioni in più al Fondo nazionale per la non autosufficienza e indire un incontro Stato-Regioni

Tornando al merito dei principi. Sono parzialmente appagata dal fatto che sostanzialmente si sia modificato il testo

cui finalità è la cura e la protezione delle persone con disabilità. In tale finalità abbiamo inserito «nel superiore interesse delle persone con disabilità grave». Ciò è importantissimo perché una delle preoccupazioni era propria quella. Vedendo al comma 3 la parola «*trust*», a molti è venuto un dubbio: qual è l'interesse prioritario? Averlo specificato al comma 2, diciamo che può tranquillizzare un po' sugli obiettivi. Aver modificato gli articoli 1 e 6 non dando esclusività al *trust*, ma aprendo ad altri tipi di investimento, credo sia una cosa positiva.

del comma 1 prevede la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Non si specificavano troppe cose e non si precisava il fatto di dover chiedere, dove possibile, il rispetto della volontà del disabile stesso o anche dei suoi genitori. Non era specificato che non fosse una priorità di questo fondo

o almeno l'accenno in una parte di questo disegno di legge, al discorso del controllo e dell'attività di vigilanza. Visto che ascoltate le cronache, sapete che è importante comunque sapere che lo Stato c'è e almeno s'impegna nella vigilanza,

non c'è alcun tipo di forzatura e temo che non si sia utilizzata un'espressione che incentivi il cambiamento. Anche i criteri di assegnazione del fondo sono contenuti in una delega e purtroppo le deleghe sono all'ordine del giorno. Spero davvero nella buona volontà delle Regioni e avrei sperato in un' azione più forte da parte del Governo, anche se il rapporto ISTAT ha

abbia risolto il problema in maniera così superficiale: lo ripeto, la spesa *pro capite*

che nella minoranza nessuna rappresentanza politica può fare il miracolo da me aspettato; quello che ho fatto, lo reputo già tale,

falsificato nei contenuti e spacciato per chissà quale soluzione. In realtà non porta a casa molto:

suo impegno. Noi componenti del Gruppo dei Conservatori e Riformisti siamo tra coloro che credevano non più procrastinabile l'adozione di un provvedimento per alleviare la sofferenza e le difficoltà di molte famiglie e la loro motivata ansia

quindi, ci riferiamo a circa 127.000 persone. Signor Presidente, tutti pensiamo che un intervento legislativo fosse necessario, tuttavia c'è chi pensa

Io invece sono convinta che non sia più sufficiente provvedere in questo modo, quando si parla e quando si interviene su temi dalla grande rilevanza sociale, come quello Le istituzioni, e quindi la politica, hanno il dovere di cambiare passo, di fare uno sforzo ulteriore per disegnare con lungimiranza gli scenari del domani, dove si intravedono già da ora chiaramente due grandi questioni: da una parte il bisogno sempre maggiore di un *welfare* efficiente e le sempre più esigue risorse disponibili, dall'altra. Si discute ancora poco in Italia - molto di più fuori dai confini nazionali

ha aperto agli italiani una finestra sulla nuova economia alla quale ci dobbiamo dedicare, sostenuta finanziariamente proprio da investimenti che debbano prevedere e contemplare la valutazione di impatto sociale.

che - magari - non avrebbero altrimenti luogo, attraverso investimenti per iniziative di imprenditorialità sociale finalizzate alla risoluzione di un problema sociale o anche ambientale.

term care*, prima citata dalla senatrice Bignami, con la conseguenza che l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi europei nell'accesso ai servizi domiciliari e residenziali, in particolare per gli anziani non autosufficienti e, più in generale, per le persone con disabilità. Il quadro generale odierno del Paese presenta un'estrema frammentarietà e disarticolazione di denominazioni di servizi, criteri valutativi, modelli di contribuzione pubblica e interventi dei Comuni. Un intervento che tenti una razionalizzazione a livello nazionale non può non rimettere fortemente in gioco la necessità di regole comuni per lo sviluppo della rete locale dei servizi, il mantenersi e aggravarsi delle diversità territoriali, non solo tra Mezzogiorno e Centro-Nord, ma anche a livello interregionale e infraregionale, a volte da Comune a Comune. Va delineato, secondo noi, un percorso di organizzazione e gestione dell'assistenza socio-sanitaria integrata da proporre in alcune realtà territoriali, ad esempio come sperimentazione di una nuova modalità di erogazione delle prestazioni essenziali esigibili dal cittadino in stato di bisogno,

Grazie non solo del "dopo di noi", ma anche di quell'assistenza alla quale tutti puntiamo, frutto di un'antica cultura di cui il Paese è portatore, ma che deve trovare una modalità moderna, in quell'integrazione socio-sanitaria

il distretto/ambito come luogo di sviluppo delle strategie e degli strumenti di integrazione, con la messa a fattor comune dei diversi attori istituzionali, pubblici e privati. La via del finanziamento partecipativo è la ricerca di soluzioni ottimali per garantire l'effettiva integrazione tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria erogate a malati cronici, malati cronici, anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con una possibile estensione ai minori con disturbi in ambito psichiatrico e ai pazienti psichiatrici, ad esempio. In un momento successivo, l'area di intervento potrebbe essere estesa ad ulteriori ambiti. I *social impact bond* sono, secondo me, lo strumento finanziario più adatto per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici a forte impatto sociale. Si tratta di un'evoluzione della finanza verso la quale dobbiamo spingere, con tutte le forze che abbiamo, per avere una finanza a sostegno degli interventi sociali, che non sono solo assistenza, ma anche un grande investimento sul capitale umano e sul futuro. Penso anche con grande speranza allo sviluppo delle società *benefit* che il nostro Governo ha voluto introdurre, tra i primi in Europa, mutuandole dal modello americano: uno strumento efficacissimo che dobbiamo saper utilizzare. Torno al merito stretto della legge in esame che, come ha già ricordato qualche collega prima di me, rappresenta uno strumento per l'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU del riconoscimento del diritto delle persone con disabilità all'autodeterminazione e a scegliere liberamente dove e con chi vivere. Si tratta copre una platea numerosa in termini assoluti (lo ricordavo prima), che però è molto ristretta rispetto al tema più ampio della disabilità. Infatti, per evidenti ragioni di copertura - deduco io - il provvedimento si concentra esclusivamente sui disabili gravi, la cui condizione non sia determinata dal naturale invecchiamento. Pur se ancora molto doveva e dovrà essere fatto, questa legge, nel testo che oggi stiamo votando, ha il pregio di introdurre una vera e forse unica novità: la disciplina dell'istituto del *trust* per fini assistenziali. Pensiamo, in particolare ai minori, per i quali i genitori spesso non possono immaginare un futuro dignitoso. Il *trust* è un istituto poco conosciuto e poco applicato a causa della mancanza di una normativa nazionale che risolva i problemi di compatibilità con il nostro ordinamento; da oggi rappresenterà una possibilità nuova per coloro che vogliono scegliere come e da chi sarà gestito il futuro del proprio caro, fornendo loro una tranquillità e una serenità che nessun altro istituto giuridico italiano consente. Concludo, signor Presidente, parlando delle risorse messe in campo, perché non c'è una buona legge senza adeguate risorse. Questo è un punto di partenza, ma tutti abbiamo riconosciuto che non sono sufficienti. Il mio Gruppo, con la senatrice Bignami, con la quale abbiamo condiviso tutti gli emendamenti, ne aveva presentato uno volto ad alimentare il Fondo con la possibilità per i cittadini di destinare allo stesso, in sede di denuncia dei redditi, l'otto per mille, rendicontando annualmente al Parlamento l'andamento della raccolta e soprattutto dell'impiego. Sono contenta che il senatore Candiani ne abbia condiviso lo spirito, sottoscrivendolo insieme a noi. Signor Presidente, noi Conservatori e Riformisti, votando favorevolmente questo disegno di legge, promettendo la massima attenzione anche su tutti i decreti attuativi che stabiliranno veramente la buona riuscita o no degli obiettivi di tutela, invitiamo però a fare di più e a gettare noi, insieme a quelle famiglie, il cuore oltre l'ostacolo.

Legge buona o legge non buona? Le casistiche sono infinite, le disabilità sono le più svariate, a seconda dei

si mettevano le cose buone su un piatto e le cose non buone sull'altro, e se tutto sommato le cose buone prevalevano sulle meno buone,

vivono una missione: vivono in funzione di questi figli che hanno totale necessità dell'assistenza dei propri genitori.

tutto ciò che è stato buttato sul campo e ne ha saputo fare una sintesi in questo provvedimento.

le piccole divergenze - che chi non ha genitori con un patrimonio debba essere abbandonato. Sgombriamo il campo da questa idea, perché forse qualcuno in tal senso ha mal interpretato. Anche noi avremmo voluto dare risposte a tutti a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il problema successivo nasce dalla terminologia: disabili gravi.

piacere sentire che la collega Bignami, che è stata molto critica e che conosce molto meglio di tanti di noi la materia, alla fine abbia dato un giudizio

concludo dicendo che anche come Lega avremmo voluto avere una legge più ampia che avesse potuto dare risposte a una platea maggiore. Però, per le ragioni che abbiamo appena

MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare, conosciuto dalla pubblica opinione come il "dopo di noi", è certamente caratterizzato - come è stato ampiamente dimostrato dal dibattito migliorativo svolto in Commissione e poi qui in Aula da un interesse e da una condivisione trasversale che si estendono ed abbracciano praticamente tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Il lavoro ha l'obiettivo di realizzare quello che viene definito come il diritto alla solidarietà,

questo provvedimento vedrà incrementate le tutele e consolidati i diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite Soprattutto si realizza la funzione di quella Repubblica di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione che ha il compito di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Da una recente indagine dell'ISTAT svolta in merito, nel nostro Paese vivono circa 3.200.000 persone con disabilità, e di queste circa 600.000 nella fascia di età da zero a sessantaquattro anni hanno una disabilità grave certificata ai sensi della legge n. 104 che regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Di queste donne e di questi uomini e ragazzi, 260.000 vivono in famiglia con i genitori o i fratelli che per questi nostri concittadini sono, per tutta la durata della loro esistenza, la principale fonte di sostegno e di assistenza. È infatti proprio la famiglia a garantire, nella generalità dei casi, la necessaria assistenza alla persona con disabilità, e spesso lo fa a costo di enormi conseguenza anche del fatto che in molti casi i servizi sociali prestati dal "pubblico", dal nostro *welfare*, non sono idonei, anzi, sono fortemente insufficienti a soddisfare le particolari esigenze di chi è affetto da grave disabilità. A questo si aggiunga lo stato di motivata angoscia e profonda apprensione dei familiari dei disabili non autosufficienti, che vivono nel costante dilemma del futuro che aspetta il loro congiunto quando un giorno non ci saranno più loro ad assisterli. non sono rari i casi, anche conseguenti al periodo di crisi economica che abbiamo attraversato nell'ultimo decennio, in cui le sostanze economiche della famiglia diminuiscono, soprattutto a causa del costo delle cure e non sono più sufficienti ad assicurare la necessaria assistenza ai loro cari. La problematica è pertanto tangibile e noi intendiamo, ove possibile, provare a restituire un sorriso ed un pizzico di tranquillità in più a migliaia di queste famiglie. Sul tema della disabilità purtroppo l'Italia parte da un forte ritardo, da una cronica mancanza di attenzione verso una riforma del *welfare* che tenga conto dell'attuale struttura sociale, delle esigenze di cura e benessere, molto diverse rispetto a qualche decennio fa e da zona a zona del nostro Paese. Il modello di *welfare* italiano, incentrato sulla delega alle famiglie, è in profonda crisi ora che i mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, frutto di anni di gestazione, arriva sicuramente ridimensionato, specialmente nella sua dotazione di risorse. Il contributo che lo Stato mette a disposizione per questa legge è di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Ritengo comunque che il provvedimento in esame abbia al suo interno aspetti molto positivi che finalmente danno risposte - in gran parte - alle domande che da sempre ci vengono poste dalle famiglie interessate al problema: quello di evitare l'istituzionalizzazione dei disabili nel momento in cui resteranno soli per la mancanza dei genitori, di aumentare la loro protezione attraverso regimi fiscali agevolati per la disabilità, di dar vita a percorsi per l'indipendenza degli individui portatori di *handicap* seri, di creare occasioni e possibilità reali di inserimento lavorativo, case famiglia, comunità, coabitazioni di disabili in appartamenti a loro dedicati, per evitare casi di segregazione, di esclusione e di diseguaglianza. Un altro obiettivo fondamentale è quello di istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni IRPEF e di prevedere agevolazioni tributarie per i *trust*. Forse non è ancora il massimo che si poteva fare, se si considera che i Comuni spendono all'incirca 7 miliardi di euro per la disabilità in generale e circa 1,5 miliardi per i disabili di cui stiamo parlando nel provvedimento. Certo le cifre che si annunciavano all'inizio del provvedimento erano molto più ambiziose, ma di fatto si sono ristrette considerevolmente. Peccato. È un'occasione in parte perduta che poteva essere utilizzata meglio da parte della maggioranza e del Governo. Il provvedimento è, senza dubbio, un segnale di speranza per le migliaia di famiglie interessate dal problema, che si traduce in attenzione concreta per tutti coloro che giornalmente si confrontano e vivono la disabilità e che devono, senza ulteriori ritardi, sentire il legislatore vicino e partecipe alle proprie esigenze, con misure concrete, pratiche e di buonsenso. Forse si poteva fare di più: è una frase fatta. Occorre, forse, fare di più con più coraggio, ma probabilmente questa che ci apprestiamo a votare oggi, con il miglioramento apportato in Senato, è la migliore soluzione possibile, nonostante tutto. Mi auguro però che non resti un provvedimento isolato: è un inizio, sì soltanto l'inizio di un percorso. Sicuramente il problema della disabilità e quello degli anziani anche non autosufficienti e di tutte le non autosufficienze presenti nelle società occidentali e nel nostro Paese si amplierà sempre più nel corso degli anni, dato che è aumentata l'aspettativa di vita. Saranno ovviamente sempre di più i problemi all'ordine del giorno. Il testo in esame rappresenta quindi certamente un punto di partenza importante. Andranno reperiti altri fondi, ancor di più di quanti ne siano stati individuati finora, che serviranno per garantire una migliore qualità della vita non soltanto ai soggetti direttamente interessati, ma anche alle loro famiglie impegnate quotidianamente in prove di vita pesantissime. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. (MpA))*. Signor Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento a me molto caro, che fa seguito ad una battaglia che ho portato avanti già nella scorsa legislatura in Commissione affari sociali

non ha visto la luce perché l'allora governo Monti non aveva dato la copertura finanziaria. Questo oggi mi fa pensare ancora di più che

demorso. Anche questo è compito di un parlamentare: non demordere, non abbandonare mai le proprie convinzioni, che devono essere portate avanti con sempre maggiore determinazione. Infatti, ho ripresentato il disegno di legge non appena varcato l'ingresso del Senato, il 25 marzo 2013.

nel mio c'era l'aggiunta virgolettata «Dopo di noi». Quello che ci apprestiamo a votare oggi è un punto di partenza importante,

il nostro percorso. È la prima volta che si fa un intervento di questo tipo da 17 legislature a questa parte, soprattutto in un Paese che ha l'ambizione di assicurare ai suoi cittadini tutti i servizi sanitari, ma anche molti servizi di carattere sociale. I numeri sono eloquenti, ce li dobbiamo dire, in Italia ci sono 260.000 persone con disabilità gravi che vivono con uno o entrambi i genitori, e tra questi circa un terzo sono genitori anziani. Il 64 per cento dei figli con disabilità grave (circa 170.000) sopravvivrà a genitori e a fratelli.

Il nuovo testo approvato alla Camera con l'assorbimento di disegni di legge *bipartisan* - del Partito Democratico, di Area Popolare, di Sinistra Italiana - ha arricchito la mia proposta, lasciandone saldi, però, i principi, il filo conduttore: tra tutti, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Il testo prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare o perché sono venuti a mancare i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Viene istituito un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinato in particolare ad attivare programmi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa la scienza si deve occupare anche di loro e le nuove scoperte scientifiche devono essere anche a loro appannaggio, al fine di impedire l'isolamento di persone con disabilità. Sono previste agevolazioni tributarie per i *trust*, nome che prendiamo dall'istituto del sistema giuridico anglosassone, che vuol dire fiducia, fido, ovvero lo strumento giuridico per la gestione di patrimoni costituiti di patrimoni costituiti in favore di persone con disabilità grave e per le famiglie con parenti disabili gravi. Finalmente un *trust* non per evadere le tasse ma per un fine nobile. La casa, ad esempio, è una delle preoccupazioni maggiori

che si prenderà cura di loro. A meno che non vengano scelti di proposito, quindi, si potrà andare oltre i nosocomi o le residenze sanitarie assistite e si andrà verso la civiltà. Già nella scorsa legislatura, come ho detto all'inizio, quella sul «dopo di noi» fu una battaglia, come si ama definirla in ambito politico*, bipartisan*. non fui il solo autore della proposta di legge che ho presentato, ma era coinvolta anche la capogruppo del Partito Democratico, Livia Turco, che voglio ricordare perché con lei ho scritto il testo che poi ho presentato all'inizio della legislatura; anche lei aveva molto a cuore questa proposta di legge.

Sono consapevole che il provvedimento sia ancora perfettibile e che non tutto è stato fatto, ma fino ad oggi, come ho già detto, nessuna delle legislature precedenti ha fatto quello che stiamo facendo noi ed è per questo che ne dobbiamo andare fieri. Sono altrettanto consapevole che da oggi, con questa legge, tante famiglie, tanti genitori, tanti figli vivranno una vita più tranquilla, certo improntata alla cura e all'assistenza di propri cari in difficoltà, ma senza l'incessante paura per il domani. È una legge di misericordia e la andiamo ad approvare nel Giubileo della Misericordia: questo accostamento mi sembra molto attinente. Il pensiero del "dopo di noi" non assillerà più tanti genitori, fratelli o parenti prossimi, rendendoli disperati, ma li conforterà il fatto che da oggi potranno scegliere. Il destino non è più uno solo, ma vi è un domani e il domani sarà sicuramente garantito. Vedete, cari colleghi, è in giornate come queste che la politica decide di dare spazio alla sua sfaccettatura migliore. E, infatti, è la politica nobile che prevale e solo i movimenti antipolitica si smarcano; ed è proprio qui la differenza, perché davanti alle necessità, ai bisogni e ai diritti dei cittadini non vi è colore politico. Insieme si trovano le soluzioni che rendono questo Paese migliore, come accaduto qualche giorno

Gruppo nato proprio sulle riforme (e questa noi la consideriamo come un ulteriore tassello della nostra finalità): siamo un Gruppo nato per le riforme, questa è una riforma sociale sulle disabilità e quindi andiamo fieri

Signor Presidente, colleghi, farò un intervento molto breve ma doveroso, visto il tema delicato e importante di questo provvedimento. In discussione generale e, oggi, in dichiarazione di voto sono già stati toccati e descritti tutti i temi

la mia considerazione è: stiamo attenti, soprattutto adesso, in periodo di riforme costituzionali, a dire che centralizzare è meglio e che sarà un vantaggio per il Paese. In questo caso, infatti, la

ai livelli del *welfare* del Nord Europa. Quindi il mio auspicio è che tutto ciò che è stato fatto da parte delle Regioni vada ad essere

una malattia che in queste Aule parlamentari ormai siamo abituati a vedere, quella dell'"annuncite". A leggere il titolo e ad ascoltare alcune relazioni e alcuni interventi siamo stati tutti portati a pensare che si trattasse di una legge quadro sulla disabilità, il cui obiettivo principale fosse quello di rifinanziare il Fondo sociale e il Fondo per le non autosufficienze, proprio quel Fondo che in questi anni i "Governi Tremonti, Sacconi e Monti" hanno praticamente prosciugato, mentre le vostre leggi di stabilità non contribuivano a migliorare la situazione.

questi tagli immettendo risorse immediate. Invece, nell'"annuncite" caratterizzante questa maggioranza,

Non viene presa in considerazione solo la mancanza di entrambi i genitori, ma anche l'incapacità o meglio la difficoltà a fornire adeguato sostegno genitoriale, dimenticando che il ruolo dei genitori è soprattutto fatto di supporto affettivo, psicologico, di sostegno di sostegno e di vigilanza e non è soltanto di tipo economico, che pure è molto importante. Si sancisce di fatto che la responsabilità dell'assistenza di una persona con disabilità grave è dei genitori e non del servizio pubblico; questo è il punto che viene messo in evidenza con questo disegno di legge. Si mette in un angolo la cultura del ruolo del pubblico, per aprire ad una privatizzazione del *welfare* che rompe con il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione. Non è un caso che si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni sociali, ma solo nei limiti delle risorse disponibili. Se si vincola tutto alla sostenibilità economica e non alla sostenibilità tra domanda e offerta, che prevede l'esigibilità di un diritto, si va nella direzione di favorire le strutture piuttosto che progetti individuali domiciliari. Nel progetto individualizzato di vita, i bisogni delle persone sono differenti e non possono corrispondere a *standard*. Questa ipotesi sarebbe possibile se si parlasse di prestazioni all'interno di strutture dove i percorsi vengono standardizzati e non costruiti in base alla persona, alla sua volontà, ma in base alla tipologia o alla gravità. Si prevedono interventi per la permanenza temporanea in soluzione abitative extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza (e grazie a un emendamento approvato ieri, non lo si può fare senza il coinvolgimento della volontà del disabile). Le situazioni di emergenza in una famiglia con disabile possono essere varie e frequenti (perdita del lavoro, malattia di un congiunto, una gamba rotta, un ricovero o anche una situazione più bella, come una nuova gravidanza e l'arrivo di un neonato) e i servizi sociali dovrebbero essere in grado di garantire ore di assistenza e risorse per proseguire l'assistenza domiciliare. Questo non è però garantito. I fondi infatti sono vincolati dalla disponibilità di bilancio, non sono strutturali e dipendono dalla sensibilità dell'amministratore di turno. L'unica alternativa percorribile sarà quindi l'inserimento della persona con disabilità in una «struttura extrafamiliare», quasi come «una cosa ingombrante», perché la struttura, vista l'emergenza, sarà la prima disponibile e non la più idonea. Sarebbe stato importante creare un reale supporto alle famiglie e alle persone in condizioni di emergenza, sarebbe stato più opportuno inserire l'obbligo di tentare prioritariamente una permanenza a livello domiciliare proprio per prevenire l'istituzionalizzazione. Anche se non è detto esplicitamente, questo disegno di legge ha come obiettivo finanziare le strutture, in quanto in nessuna parte di questo provvedimento si parla di assistenza domiciliare. E questa è una delle più grandi richieste che fanno le famiglie. Il diritto al "dopo di noi" deve essere garantito per tutti. E il *trust* non è per tutti. Nel momento in cui si fa riferimento a beni o a patrimoni trasferiti ad assicurazioni, banche o fondazioni grazie all'utilizzo del *trust*, si escludono i disabili che vivono in famiglie a basso reddito. Esiste allora una sproporzione tra quanto viene destinato ai programmi per tutti i cittadini disabili chi ha potenzialità economiche tali da consentirgli di stipulare un *trust*, che appunto è un accordo basato sulle finanze, attraverso cui le famiglie lasciano i patrimoni a fondazioni, istituti e privati che gestiranno le loro vite. È evidente come il *trust* non sia una soluzione per tutti e come accresca la forbice sociale tra i ricchi e i poveri non prendendo pienamente in considerazione l'autodeterminazione del disabile.

comporta un forte impoverimento dei territori, del *welfare* pubblico dei territori, proprio di quegli enti locali e di quei servizi socio sanitari pubblici che denunciano da anni la mancanza di risorse e l'impossibilità di garantire assistenza vera. Il tema quindi sarebbe dovuto essere come aumentare le risorse pubbliche a sostegno del *welfare* pubblico. Anche questo è un tema che avete rimandato *(Applausi delle senatrici politica di questo Governo e di questa maggioranza. Per questo motivo il voto di Sinistra Italiana sarà un voto di astensione. *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatori, questo disegno di legge dà risposta a bisogni reali percepiti nella nostra società. Si stima che il 15 per cento delle famiglie, prime e fondamentali istituzioni assistenziali italiane, sia interessato da casi di disabilità. Per il disabile grave la vita con i genitori può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali, ma occorre dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio a carico dei componenti. Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano. Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante, il dialogo tra le famiglie da una parte e i servizi dello Stato dall'altra è l'incertezza del "dopo": "dopo" la nascita di un bambino disabile, "dopo" la scuola, "dopo" la formazione, "dopo" la morte dei genitori. di non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare, spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonistico con i servizi. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali, che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative. Molte delle associazioni ascoltate, nel corso delle audizioni svolte in Commissione, hanno ribadito fortemente il concetto che la grande sfida non è solo quella di affrontare le emergenze quotidiane, ma di garantire ad ogni persona disabile il diritto a una vita dignitosa, indipendentemente dal sostegno dei familiari. Il provvedimento al nostro esame ha appunto il proposito di passare da una logica meramente assistenziale alla garanzia di diritti individuali inalienabili. Di fatto, i riferimenti costanti alla nostra Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, soprattutto alla Convenzione ONU, nel suo articolato molto preciso e dettagliato, ci aiutano a mettere a fuoco il cambio di passo che questa legge rende necessario e indifferibile. Ci permettono di capire perché non si può fare un passaggio alla semplice inclusione sociale, senza mettere in gioco quella che è una vera e propria integrazione. Si tratta di una legge giusta e necessaria, arrivata finalmente dopo anni di tagli ai servizi sociali, alle politiche sociali, ai servizi alle famiglie, soprattutto a quelle in forte difficoltà, quali quelle con figli disabili gravi. Il lavoro svolto in Commissione è stato altamente costruttivo: maggioranza e opposizione si sono costantemente confrontate non per rallentarne i lavori, considerato anche il cospicuo numero degli emendamenti presentati, ma per legiferare, ai fini di un adeguamento del progetto di vita individuale, in direzione della deistituzionalizzazione, in coerenza con i principi della citata Convenzione ONU. Uno dei meriti maggiori di questa legge è proprio quello di aver rilanciato una nuova alleanza tra Stato e famiglia, un nuovo *welfare*, grazie ad una sinergia del tutto innovativa tra pubblico e privato: fondo pubblico, *trust*, fondazioni senza scopo di lucro, sussidiarietà orizzontale e verticale che dialogano tra di loro. Lo Stato e le Regioni che si avvicinano a tutti, ricchi e meno ricchi, con una ridotta istituzionalizzazione e più autonomia di scelta tra le diverse forme di vita a misura familiare. un approccio che mira a creare una sinergia che non solo valorizza le risorse esistenti, rese disponibili dallo Stato e dalla famiglia, ma le moltiplica e le reinveste, con un solo obiettivo specifico: garantire migliori condizioni di vita ai figli disabili e a quanti versano in condizioni analoghe. Il provvedimento in esame, infatti, si ispira anche a quella solidarietà orizzontale che crea relazioni virtuose tra le famiglie delle persone disabili, immaginando un sottile legame di collaborazione e di integrazione tra di loro. Questo approccio ha permesso di mettere le persone e non le categorie al centro dell'attenzione: il dibattito - lo voglio ribadire - si è sempre concentrato sul benessere del singolo, sulla pluralità delle problematiche dei singoli, sul rispetto dei loro diritti, che finora non erano stati garantiti. Il cuore del provvedimento è l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e ai disabili prive del sostegno familiare, al quale è possibile accedere con alcuni requisiti.

Le risorse che lo Stato trasmette alle Regioni vanno destinate a progetti flessibili, in costante evoluzione e fortemente personalizzati. La personalizzazione dei progetti include, oltre all'adeguata assistenza sul piano sociale, anche un approccio tecnologicamente sofisticato, alla luce delle nuove possibilità che si dischiudono per facilitare nuovi possibili livelli di autonomia.

del maggior livello di autonomia possibile ai disabili senza assistenza. Dobbiamo superare l'erogazione anonima di prestazioni omogenee, uguali per tutti, per affrontare i bisogni di disabili che, invece, sono profondamente diversi tra loro. Ogni persona deve rimanere se stessa, con il suo stile di vita, analogo a quello che aveva nella sua famiglia, garantito da una continuità di cure e attenzioni sul piano sociale, oltre che assistenziale. Per questo, occorre attivare programmi di supporto alla domiciliarità, impedendo l'isolamento dei disabili e utilizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. in esame guarda con particolare attenzione alla possibilità di realizzare interventi di residenzialità tesi a creare strutture alloggiative familiari e, per questo, possono prevedere oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e anche di attrezzature. Nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versate per rischi di morte. Si prevede, inoltre, che i trasferimenti di beni e di diritti a causa di decesso, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* siano esenti dall'imposta di successione e donazione, purché il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile. alcuni si è sostenuto che le misure contenute nel provvedimento in esame non sono sufficienti e che sarebbe stato necessario fare di più. Certamente il disegno di legge, come ogni altro, è perfettibile. Per questo, le giuste proposte di allargamento della platea, di riconoscimento di nuovi diritti alle famiglie e di maggior stanziamento delle risorse dovranno rappresentare le direttive da seguire per i futuri interventi in materia. Ad esempio, è stata immaginata una misura grazie alla quale l'assistenza dei genitori ai figli gravemente disabili venga computata, in termini di durata, nel tempo necessario per andare in pensione, in considerazione del fatto che l'assistenza continuativa a soggetti gravemente disabili è effettivamente usurante per le famiglie. Gli effetti concreti che il provvedimento in esame sarà in grado di produrre nel prossimo futuro dovranno essere valutati costantemente ed attentamente in termini di efficacia ed efficienza, al fine di correggere eventuali disposizioni inadeguate, incentivare le pratiche più positive ed introdurre nuovi meccanismi di sostegno alle persone disabili. Voglio ringraziare pubblicamente la relatrice, senatrice Parente, che non ha mai abbassato la guardia, né rallentato l'attenzione sulla necessità di fare una buona legge «presto e bene», come soleva spesso dire durante il dibattito (cosa che, a nostro avviso, è stata compiutamente realizzata). Presto e bene vuol dire dare risposte concrete a bisogni urgenti, a situazioni di emergenza e a voci di sofferenza. Quello che ci accingiamo a votare è, dunque, un disegno di legge che si fa carico delle difficoltà delle persone disabili e delle loro famiglie; che, dopo troppi anni di tagli e disinteresse, interviene in positivo con un'operazione sistematica di progettualità assistenziale e di garanzia dei diritti. Per questi motivi, annuncio il voto convintamene favorevole del Gruppo Area Popolare.

è la prima volta che mi capita dall'inizio della legislatura di trovarmi di fronte ad un disegno di legge che è stato denunciato al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. A coinvolgere tale organismo è stato il Coordinamento sanità e assistenza (CSA) fra i movimenti di base, che opera ininterrottamente dal 1970 a favore dei diritti delle persone che non possono difendersi da sé. Il CSA e la Fondazione promozione sociale ONLUS avevano segnalato per tempo con allarme e vivissima preoccupazione il carattere illegittimo e ingannevole di tale proposta di legge. Tant'è che avevano anche inviato una lettera aperta intitolata «Gravissima proposta di legge sul "dopo di noi": ignorate le leggi vigenti per le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia e concreto rischio di iniziative clientelari».

Ciò stride vistosamente con quanto denunciato, specialmente se viene citata la sussidiarietà orizzontale e la collaborazione proficua tra pubblico e privato. privato. Questo atto, l'ennesimo in questa legislatura, pensiamo sia palesemente affrontato per soddisfare clientele e appetiti privati. Il disegno di legge sul "dopo di noi" non nasce dunque nel migliore dei modi. Al Senato la relatrice ha apportato delle migliorie, ma senza incidere nella sostanza. Già nel titolo si legge: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare». Intento nobile, ma che già crea una disparità tra disabili gravi e non; e avete insistito all'inverosimile ad aggiungere il termine «grave», in un ambito dove assolutamente si dovrebbe evitare di fare discriminazioni di sorta. M5S)*. È chiaro come la gestione della vita dei disabili sia sempre più delegata al privato, mentre lo Stato è depotenziato, assumendo un ruolo di comparsa: questa è una inversione dei ruoli per noi inaccettabile. All'interno del disegno di legge si parla di istituire un *trust*, una figura giuridica di un altro ordinamento che viene proiettata nel sistema italiano, quasi fosse possibile fare un mero copia-incolla da un ordinamento all'altro, senza considerare le diversità e le specificità di ogni Nazione. Ogni Paese ha le sue regole, tradizioni e livelli diversi di assistenza. Nell'elaborazione di un disegno di legge che, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe agevolare e migliorare le condizioni dei disabili, avremmo voluto vedere meno approssimazione. Il *drafting* legislativo e le regole della *better* *regulation* seguono criteri lineari e una progettualità che qui non vediamo. L'*iter* è stato lungo e tortuoso e la relatrice ha presentato ben tre emendamenti

creando un vuoto normativo molto grave, secondo noi. Facciamo notare che nella prima stesura del testo alla Camera non era stato preso in considerazione il *trust*, inserito in un secondo momento. Ma come si è arrivati a introdurre questo strumento?

e dopo che l'associazione "Il trust in Italia" si è pronunciata attraverso il suo vice presidente Maurizio Lupoi che, stando a quanto si legge sui giornali, è il vero estensore della legge. Già solo per questo riteniamo che questa parte del disegno di legge vada abrogata *in toto*. Inserire in un disegno di legge dedicato alle persone disabili uno strumento che andrebbe normato e regolato con infinita cura e attenzione è l'ennesima forzatura legislativa. La parola *trust* si traduce in italiano con il termine «fiducia», ed è proprio questa che le persone in difficoltà abbisognano: una forma di fiducia e garanzia universale garantita dallo Stato per tutti i cittadini e non solo per coloro che si possono garantire, in quanto facoltosi, privilegi o favoritismi di sorta. Si è anche sentito chiaramente nell'audizione che persone con gravi disabilità,

chi giova quindi questo istituto? Si fanno veramente gli interessi della persona disabile o si favoriscono gli intermediari privati? Se l'interesse dei proponenti fosse stato autenticamente quello di tutelare i disabili, si sarebbe intervenuti valorizzando le strutture esistenti e migliorando in generale i livelli di assistenza, magari iniziando dalla scuola e fornendo un adeguato sostegno ai ragazzi, anziché tagliare sugli insegnanti di sostegno. Così il progetto è chiaro. Si tagliano i fondi pubblici già esigui di per sé, si creano conseguentemente situazioni di inefficienza e poi arriva la maggioranza con la soluzione: si crea un *trust* dove si mettono dentro fondazioni bancarie e soggetti privati, ONLUS e cooperative, che molto probabilmente si tingeranno di un festante rosso.

si trovano nella disperazione che, ogni anno, provoca suicidi, annientamenti di interi nuclei familiari, isolamento e segregazione di genitori che, da anziani, non hanno la certezza di che fine farà il proprio figlio. Troppo deboli sono state le indicazioni di principio. In pratica, c'è un'annacquata indicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Avevamo proposto che il provvedimento fosse coerente come da articolo 19 della Convenzione ONU, in particolare all'assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite progetti veramente personalizzati e *budget* destinati direttamente alle persone in questione da poter investire in assistenti personali liberamente scelti e formati con l'aiuto degli amministratori di sostegno. Questo disegno di legge, invece, propone una direzione unica per le persone che vivono oggi con le famiglie, costringendole in un futuro a vivere in strutture gestite da terzi. Il "dopo di noi" diviene a questo punto un capitolo di spesa, un fondo, l'ennesimo, con l'ennesimo decreto di riparto e gli stessi interventi regionali, più o meno adeguati a seconda se vivi al Nord o al Sud. Qui devi essere fortunato perché, se vivi al Sud, sei sfigato in partenza. Notiamo che, mentre nel disegno di legge n. 2232 sono molto lucidi i passaggi che trattano del fondo e del *trust*, restano fumose o si rimandano le parti concernenti la definizione dei livelli assistenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare che, a loro volta, si rimandano a un decreto che si dovrà varare entro sei mesi dall'entrata dall'entrata in vigore di questa legge. Facciamo presente, a proposito dei riferimenti ai limiti delle risorse disponibili, che esiste la sentenza della Corte costituzionale n. 509 del 2000 che ha evidenziato che, secondo un principio desumibile della giurisprudenza della stessa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito a ogni persona come costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti. Il bilanciamento, tra l'altro, deve tener conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone. Dunque, sulla base della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, le Regioni e le ASL devono «in ogni caso» garantire il nucleo irriducibile del diritto alla salute» stabilito

All'articolo 5, in sostanza, si ingrassano le assicurazioni private, creando ammanchi ai fondi pubblici. In questo articolo si parla delle detraibilità possibili su polizze assicurative stipulate con la finalità di tutelare le persone a noi care che hanno disabilità. In questi giorni è pervenuta una lettera al Presidente della Repubblica da parte di familiari di disabili, nella quale si ribadisce il concetto che questo disegno di legge non risponde ai cittadini e ai loro bisogni, con la preghiera di non firmarlo. La loro alternativa, da noi condivisa, è stabilire che le risorse previste nella legge di stabilità

meglio i nostri concittadini. Chissà se il legislatore sì è accorto che in questo Paese le fasce di povertà sono in aumento e la forbice tra il ricco e il povero è sempre più marcata! Questo modo sbagliato di gestire il *welfare* è il vero artefice di tanta disperazione. Il dolore più grande per una persona è non sopravvivere al figlio. Ma forse ce n'è uno ancora più lacerante: desiderare in modo inconfessabile che il figlio disabile possa col genitore finire la propria esistenza, dramma che pesa come un macigno nella coscienza collettiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge al nostro esame affronta una questione di grande importanza: fornire un supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. questo che ha registrato una sensibilità trasversale, come abbiamo visto dal numero e dalla profondità - se mi consentite - degli interventi svolti in quest'Aula. Certamente l'esame del testo riscontra una maggiore consapevolezza in chi abbia conoscenza diretta della disabilità. Ma anche chi non avesse una esperienza personale, è rimasto certamente colpito dalle immagini della cronaca, che mostravano esseri umani maltrattati e umiliati nella propria dignità, in cosiddette case di cura o sedicenti centri di riabilitazione. Credo profondamente che la politica, prima ancora della legge, debba dare le risposte più adeguate affinché non abbiano mai più a ripetersi questi episodi criminali. il disegno di legge in esame mette in campo talune giuste proposte ad alcune di dette questioni, e lo fa ponendo al centro il disabile e la sua famiglia; lo fa quando parla della possibilità di pensare al futuro costruendo un percorso che contempli non l'istituzionalizzazione, ma la possibilità di poter costruire la propria vita come un abito su misura; lo fa dando serenità ai genitori nel durante noi e la certezza di aver assicurato la miglior soluzione al dopo di noi.

Ricordo - come hanno già fatto altri colleghi - che nel biennio 2012-2013, in Italia, sono 3,2 milioni le persone con disabilità, indicate dall'ISTAT con la nuova definizione di «persone con limitazioni funzionali». La materia è ancora largamente regolata dalla legge n. 104 del 1992 e bisogna registrare che permangono termini difformi nelle definizioni utilizzate nel complesso ambito legislativo sinora maturato. legge al nostro esame, dopo l'approvazione della Camera, dove dovrà tornare per l'approvazione definitiva, contiene - a mio parere - delle apprezzabili modifiche che abbiamo introdotto in Commissione lavoro del Senato. Nel merito del provvedimento abbiamo espresso la ulteriore preoccupazione che, dalla disciplina oggetto di intervento, possano rimanere esclusi alcuni soggetti, molto deboli, che pure sono meritevoli di tutela, anche se non rientrano nella definizione di disabile grave. La straziante preoccupazione dei genitori è quella che, dopo di loro, nessuno possa prendersi cura dei propri cari. Ovviamente, questo comporta il reperimento di risorse finanziare, che si devono rintracciare nell'ambito del bilancio dello Stato, se si vuole fare fronte a una problematica così rilevante. Il riferimento alle disabilità gravi - richiamato nelle disposizioni al nostro esame - è appunto all'articolo 3, comma 3, della legge-quadro, che definisce come disabile grave la persona che, a causa di «minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione». tuttavia disabilità, in forma apparentemente minore, che segnano la vita non solo delle persone che le vivono, ma anche delle loro famiglie e, spesso, di intere piccole comunità. La necessità di una integrazione alla legge quadro, che ha più di venti anni di vita, nasce anche dai continui casi di cronaca che ci hanno costretto a leggere di persone a libertà limitata. È fondamentale evitare che persone con disabilità possano essere escluse o marginalizzate, con il reale rischio che per loro il dopo di noi significhi istituzionalizzazione e quindi un evidente peggioramento della propria qualità di vita. È nostro preciso dovere garantire il diritto a ciascun individuo disabile di vivere dignitosamente, anche senza la propria famiglia di origine, senza subire, una volta fuori dalla propria casa, isolamenti o trattamenti che hanno poco di umano. In tal senso la normativa che stiamo per approvare propone una protezione dell'individuo e del suo patrimonio, per realizzare il più compiutamente possibile la sua libertà. Le norme sui *trust*, sui vincoli di destinazione e sui fondi speciali, così come la maggiore detraibilità per le polizze assicurative, sono assolutamente apprezzabili, ma non bastano. Sono state studiate per le famiglie che hanno comunque un patrimonio da mettere a disposizione per l'autosufficienza del proprio caro, ma non riguardano chi non possiede nulla. A questi ultimi è necessario che provveda l'intervento pubblico, che deve essere meglio articolato, e non solo per il "dopo di noi", ma anche per il "durante noi". Purtroppo le risorse sono andate gradualmente diminuendo con la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, che hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nell'affidamento di molti servizi ai disabili. Tra l'altro, l'assistenza organizzata dai Comuni registra caratteristiche estremamente differenziate sul territorio nazionale. Va quindi fatto qualcosa di più, innanzitutto per dare parità di trattamento, e quindi di dignità, a tutti i disabili, ovunque essi risiedano. È necessario, inoltre, affrontare il problema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, contemperandoli con i livelli essenziali di assistenza in ambito socio-sanitario. Ora chiediamo, quindi, lo sforzo ulteriore di non guardare solo all'oggi, ma anche al domani. Dare piena attuazione al diritto ad autodeterminare la propria esistenza alle persone con disabilità - sancito in sede internazionale - significa sopratutto consentire di scegliere come e dove vivere durante tutta tutta la propria vita, nel rispetto dei nostri valori costituzionali. L'orizzonte temporale deve essere quindi più lungo, perché deve consentire non solo l'attuazione delle norme che andiamo ad approvare oggi, ma anche il compimento delle tante iniziative messe in campo a livello territoriale, che guardano al domani e hanno necessità anche di risorse pubbliche. Prima di concludere - lo faccio con un po' di emozione - voglio raccontarvi la storia di Diego. Diego ha la mia età, è una persona affettuosa, crede nell'amicizia, si fida degli altri. Diego per una sigaretta ti apre le porte di casa, adora il suono delle campane, alla domenica le suona pure. Diego suona il pianoforte senza aver studiato la musica. Diego adora la montagna e ama la vita. Diego fino a poco tempo fa, grazie a un imprenditore illuminato, lavorava; poi, purtroppo, l'azienda è andata in crisi e ha chiuso. I genitori di Diego non si arresero e riuscirono a farlo inserire in una cooperativa sociale nell'ambito di un progetto di lavoro mirato sperimentale. Diego ogni mese ha portato con orgoglio a casa la sua busta paga, si è sentito importante; ora il progetto non c'è più e Diego ha riperso il lavoro. I genitori di Diego, che sono anziani, ogni fine mese stampano una vecchia busta paga e vi inseriscono lo stipendio con i loro risparmi. Diego, quindi, continua a essere orgoglioso di se stesso. Diego è un mio amico, ha un *deficit* intellettivo, ogni tanto la saliva gli esce dalla bocca ed è un disabile grave. Diego non potrà usufruire della legge sul dopo di noi e come lui tanti altri. A tal proposito desidero ringraziare la relatrice Parente e il sottosegretario Biondelli per aver accolto il mio ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione proprio queste situazioni. Credo che il disegno legge che a breve approveremo sia un passo in avanti importante, che accoglie l'aspettativa di tante famiglie, ma che non deve fermare il percorso di civiltà e sussidiarietà che oggi abbiamo intrapreso. Ognuno di noi deve impegnarsi a far sì che nessuno dimentichi i tanti «Diego» e le loro famiglie. Per le ragioni esposte, con la consapevolezza che molto ancora dobbiamo ai disabili e alle loro famiglie, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signora Sottosegretario, oggi è una giornata importante e bella davvero. Possiamo esserne orgogliosi. Questo provvedimento è atteso da molte persone e una di queste si chiama Annarita, che conosco da sempre. È una madre coraggio mi ha detto tante volte: «Stefania, fate presto, fate presto. Cosa accadrà a mio figlio Mario quando io non ci sarò più?». Come Annarita, altre migliaia di madri e padri vivono questo assillo e per anni hanno fatto appello alle istituzioni e alla politica, ma soltanto ora, oggi, ricevono finalmente una risposta dal Parlamento italiano. Il Partito Democratico voterà con convinzione e gioia questo disegno di legge. Livia Turco iniziò tanti anni fa un percorso e mi incoraggiò, da giovane amministratrice comunale, a farmi carico e a occuparmi del problema. Mi si è aperto un mondo, un mondo di bisogni silenziosi e dolorosi. Da allora, il percorso trova oggi finalmente un grande traguardo raggiunto. Ringrazio, quindi, tutti i colleghi che sono intervenuti, di ogni forza politica, e che hanno dato consigli e suggerimenti, che non si sono tirati indietro, chiudendosi in un mondo inconcludente e giacobino. In particolare, voglio ringraziare i colleghi della Commissione lavoro, le mie colleghe di Gruppo, senatrici Favero e D'Adda, che sono intervenute, così come gli altri colleghi e colleghe

della sottosegretario Biondelli, che ha condiviso con noi questo cammino, oggi portiamo alla votazione del Senato un testo visibilmente migliorato rispetto al lavoro, già positivo, fatto alla Camera. Ma è nel Paese, tra le famiglie, con le associazioni e le che questa norma da anni prende corpo, come ha detto bene la relatrice. Le vere protagoniste di questo provvedimento sono le famiglie, quelle specifiche famiglie. Ognuno di noi convive con la paura della morte, e ciascuno di noi pensa ai propri figli come all'eredità di vita, sperando che essi ci accompagnino fino alla fine. Per questi genitori, invece, non è così. Annarita e tanti altri sono assillati dal futuro. Il "dopo di noi" è una cosa seria e non è tema da *show*, da scandalismi o disfattismi, la risposta quasi corale del Senato la dice chiaramente lunga. Nessuno qui è esclusivo depositario del dolore di queste famiglie; nessuno ne può essere l'interprete totalitario. Noi abbiamo il dovere di dare delle risposte credibili. «Queste piaghe devono essere ascoltate», ha detto Papa Francesco. Mi è piaciuta la collega Argentin, deputata del PD, che ha detto che questo provvedimento avrà lo scopo di dare tanti sorrisi a persone che, dal momento che hanno messo al mondo un figlio, hanno vissuto il senso di colpa e il lutto di elaborare un limite che hanno creato. Cerchiamo di capirci: il "dopo di noi" è una risposta soprattutto sociale ad una platea definita, quella dei disabili gravi, ed è bene che sia così, perché le risposte devono essere diverse e specifiche. Disabili gravi sono le persone affette non solo da gravi patologie fisiche, ma anche da ritardi mentali e da gravi ritardi cognitivi che gli impediscono di scegliere il proprio futuro. E cosa fa il *trust*, da alcuni demonizzato? Crea il *trustee*, che è un garante (spesso sono fratelli e sorelle) che permetterà di supportare la volontà di chi è stato precedente a lui. È un istituto positivo, un'ulteriore possibilità.

prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Si tratta, in sostanza, di una visione utile e aperta, non statalista, più trasparente, che vede un maggiore protagonismo dei disabili e delle loro associazioni; una visione positiva della società, che è fatta in gran parte da persone competenti e generose e non sempre da delinquenti incalliti, come qualcuno vorrebbe paventare.

ad associazioni, cooperative, operatori del sociale. Questo è un provvedimento serio, finalizzato a persone specifiche, da non confondere con le altre generiche - ma certo utilissime - politiche per la non autosufficienza, da inserire anche all'interno di un disegno nuovo di politiche sociali, più strutturate e moderne, che ci ha visti protagonisti già con la riforma del terzo settore, osteggiata peraltro dagli stessi che oggi osteggiano il "dopo di noi".

quindi, dà risposte a chi, purtroppo, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti, a chi non può parlare. La legge richiama importanti convenzioni E sono proprio questi bisogni che hanno spinto il nostro impegno in Commissione lavoro, per migliorare il testo pervenuto dalla Camera. In questa sede vi è stato il grande lavoro della Commissione, della relatrice e del Governo, che ha voluto accettare e accogliere proposte importanti; così come sono stati recepiti i pareri di tutte le Commissioni, in particolare della Commissione finanze. Si mette al centro il progetto individuale con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche a evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,

migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal codice civile. Aggiunge, non toglie. Modernizza e rafforza le opportunità. Importante è aver inserito la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità, utilizzando gli articoli indicati dal codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative. Sono tanto i punti importante di questa legge, come importanti sono state le novità introdotte nell'articolo 6, che modifica

Concludo. Oltre alla gioia e all'entusiasmo, il Partito Democratico, nel votare questo importante provvedimento, sente anche tutta la responsabilità nei confronti delle persone disabili Governo, Parlamento, Regioni, enti locali, ONLUS, fondazioni, istituzioni, *trust*, volontariato e associazioni hanno ora uno strumento in più. Noi ci mettiamo testa e cuore nel dar voce ad Annarita e a tutti gli altri genitori. «non dimentichiamo che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Con queste parole ferme e dolci di Papa Francesco, annuncio il voto positivo del Gruppo del Partito Democratico su questo importante provvedimento. "Dopo di noi" non è solo assistenza, è la vita dopo mamma e papà. Salutiamo gli studenti del corso di diritto parlamentare dell'Università di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Non essendo presenti altri Vice Presidenti, per meno nobili motivi sospendo la seduta fino alle ore 11,25. *(La

Signor Presidente, ieri, con una certa, ma non eccessiva sorpresa, ho letto una nota di agenzia, secondo la quale il senatore D'Anna, della cui assenza mi dispiaccio, avrebbe affermato che le misure di sicurezza poste a protezione della senatrice Capacchione Capacchione sarebbero del tutto destituite di fondamento. Tutti noi conosciamo l'impegno profuso dalla senatrice Capacchione nel contrasto alla criminalità organizzata, in specie camorristica, nella sua precedente attività di giornalista - un contrasto non parolaio, come quello che, ahimè, da un po' di tempo è di moda, per qualche chiacchierone dell'antimafia

per dimostrare quanto ingenerose e ingiuste siano le osservazioni del senatore D'Anna. Devo però fare due osservazioni. La prima è che il senatore D'Anna è persona troppo intelligente per non comprendere come questo genere di dichiarazioni sia variamente interpretabile, in prossimità di una campagna elettorale importante, proprio in quelle terre, che per la prima volta vedono il Gruppo di A-LA sostenere il candidato del Partito Democratico. Il senatore D'Anna, peraltro, ben avrebbe potuto, essendo ormai non più clandestino l'ingresso in maggioranza del suo Gruppo politico, rivolgersi direttamente a un Ministro della sua maggioranza, il Ministro dell'interno, per chiedere conto e ragione delle misure di sicurezza. Alla senatrice Capacchione, a nome mio personale e del Gruppo, intendo manifestare la più assoluta solidarietà vorrei aggiungere invece a Rosaria Capacchione che, sia io che gli amici di Forza Italia, siamo e saremo sempre vicini a lei.

organizzata, ovvero le modalità di esecuzione delle sue attività, nell'ambito del territorio casertano,

un libro che, per essere stato scritto in quel modo, denota una conoscenza approfondita del fenomeno in quelle terre;

È evidente che un impegno del genere non può che esporre il suo autore a una condizione di attenzione da parte della criminalità organizzata. Basta soltanto prendere in considerazione quel libro per capire come chi lo ha scritto si sia esposto in maniera seria ad eventuali avversità che provengono da un determinato ambiente. Forse per questa ragione, credo che non tutti, forse neanche il senatore D'Anna, hanno avuto il piacere di leggere quelle pagine e quelle storie che Rosaria Capacchione ha scritto ed è probabilmente la mancanza di conoscenza della persona, del suo lavoro e del suo impegno che avrà indotto, forse con un minimo di superficialità, se non tanta, ad affermare

essere su piani diversi nell'ambito di un rapporto corretto e di confronto democratico non significa aggressione né da parte di taluni che aggrediscono

Per queste ragioni, invitando tutti alla sobrietà e al confronto democratico sulle varie questioni e sui contenuti dei provvedimenti che vengono di volta in volta all'esame, invito a questo tipo di moderazione. Per quanto riguarda l'affermazione finale del senatore Palma circa la possibilità per il senatore D'Anna di rivolgersi al Ministro dell'interno, devo ancora una volta precisare, ove mai non fosse bastato per il passato, che noi stiamo sostenendo questo Governo sulle riforme e su quei provvedimenti che riteniamo di poter condividere, ma non per questo riteniamo i componenti dell'attuale compagine di Governo nostre

Presidente, mi scuso se non potrò rispettare il suo invito a non fare considerazioni politiche. Ciò è davvero impossibile vista questa vicenda, che definire spiacevole è poco. Pertanto, mi scuso in anticipo se dirò qualcosa che potrà urtare qualche suscettibilità. Siccome sono napoletano e ho cominciato

prezzi durissimi. In quest'Assemblea vorrei fare qualche brevissima considerazione, perché, sinceramente, non mi basta nemmeno questo applauso, un po' peloso, se posso dire così,

politica rilevantissima, e sono stati vittima, come sappiamo, di minacce e di intimidazioni perché hanno avuto il coraggio di dire ad alta voce cose che invece altri non dicono, anche se le pensano.

non del senatore D'Anna ma del senatore Verdini. Lo dico io che, come i miei colleghi sanno, in quest'Assemblea sono uno di coloro che hanno molto da dire e da discutere sulla necessità di riformare alcuni aspetti della giustizia penale di questo Paese, che non mi convincono. sono uno di quelli che pensano che andrebbero riformati alcuni elementi che hanno a che fare con la custodia cautelare, tanto per dirne una, e che, per l'appunto, la custodia cautelare che dura troppo tempo

che l'onorevole Nicola Cosentino è vittima di una sorta di vendetta dello Stato, perché in galera da molti giorni senza processo. La seconda: che vengono candidati in alcune liste alle elezioni comunali di Napoli alcuni esponenti politici, o presunti tali, parenti di primo o secondo grado e anche omonimi di *boss* della camorra. La terza: che a Saviano e alla Capacchione bisogna togliere la scorta. Queste tre affermazioni le metto in fila, perché non sono dette in maniera casuale: sono un palese ed evidente atto politico; sono un palese ed evidente messaggio politico. E allora, signor Presidente, mi dispiace, ma a me non basta semplicemente la solidarietà postuma a Rosaria Capacchione. Il problema si pone prima: quando si fanno le liste e quando si fanno le alleanze. le alleanze. Chiunque parla di questo, dovrebbe sempre ricordare cosa è successo a Napoli e in Campania in tutti questi anni. Vorrei anche dire - e lo dico dalla tribuna del Senato a questo giovane candidato, nipote di un *boss*, che dice: «Che volete, che sarà mai! A Napoli, alla fine, siamo un po' tutti camorristi»: no, caro no, caro candidato della lista di AL-A al Comune di Napoli, a Napoli non siamo tutti camorristi. Io vengo da una storia che è la stessa di Angelo Vassallo, di Giancarlo Siani, di Mimmo Beneventano e questa cosa non l'accetto, non accetto la solidarietà pelosa

ben altro atteggiamento rispetto alla questione e quindi mi dispiace ancora una volta dirlo: altro che non fare considerazioni politiche! Io le considerazioni politiche le faccio fino in fondo, le faccio a testa alta e non ho paura di dirlo. senatore Zanda,

Sono ingiustificabili per qualsiasi ragione, politica, elettorale, di campagna elettorale, di concorrenza nel territorio, possano essere state pronunciate. sono rese molto più gravi e, quindi, vanno prese molto seriamente, perché sono riferite a due persone alle quali le autorità dello Stato, dopo aver lungamente e attentamente valutato le circostanze, hanno ritenuto giudiziariamente, giudiziariamente, per ragioni serie confermate dalle indagini, di dover assegnare una seria tutela perché possano essere difese in un territorio che tutti noi sappiamo porre in pericolo di vita tutte le persone perbene che si ribellano a un equivoco e a un difficilissimo e delicatissimo ambiente. Questo è il luogo nel quale Rosaria Capacchione e Roberto Saviano svolgono la loro attività. Voglio Voglio accogliere l'invito del presidente Calderoli, perché la fase elettorale spingerebbe anche a parlare di politica e non lo farò. chiudendo, che mi ha fatto molto piacere sapere dai diretti interessati che poco fa il senatore Verdini ha chiamato la senatrice Capacchione e le ha chiesto scusa a nome suo e del senatore D'Anna. *(CoR)*. Signor Presidente, credo che il collega D'Anna non abbia brillato per eleganza e correttezza di rapporti parlamentari. che, attraverso le scuse formulate alla collega Capacchione per il tramite del senatore Verdini, i rapporti che si addicono tra colleghi in questa Assemblea sono stati ripristinati.

Sulla base della lettura del libro di Rosaria Capacchione, Vincenzo D'Anna avrebbe potuto chiedere scusa direttamente e, magari, mandare un mazzo di fiori a Rosaria Capacchione e concludere l'incidente. Sono napoletano e, a differenza dell'amico De Cristofaro, non penso sia questa né la sede, né l'occasione per svolgere la campagna elettorale sui candidati al Comune. Credo che l'insinuazione del senatore D'Anna fosse impropria dal punto di vista del codice parlamentare. essere in maggioranza, essere all'opposizione, essere né in maggioranza né all'opposizione, come legittimamente il collega Falanga rivendica per il Gruppo AL-A, non significa avere una corsia privilegiata per l'esercizio del sindacato ispettivo. Signor Presidente, più volte, da parte di tantissimi colleghi, abbiamo fatto presente che c'è sciatteria e disattenzione da parte del Governo di fronte al nostro esercizio di sindacato ispettivo. la risposta alle interrogazioni avesse un ritmo diverso a seconda se sediamo tra i banchi della maggioranza o quelli dell'opposizione, sarebbe un'offesa al Parlamento ancora più sgradevole di quella fatta dalle insinuazioni sul privilegio - non so se negativo o positivo, ma non è un privilegio essendo dettato da condizioni di sicurezza - della scorta per una collega che ho sempre visto esercitare con grande impegno e serietà sia il mestiere di giornalista, sia il non mestiere di mandato parlamentare, che non legittima

il Movimento 5 Stelle, naturalmente, si associa alla manifestazione di solidarietà alla collega Capacchione e certamente anche a Roberto Saviano. stigmatizziamo fortemente le dichiarazioni del senatore D'Anna che, una volta ancora, ha gettato discredito, primariamente su se stesso ma, indirettamente, sull'intera istituzione che noi tutti ci troviamo qui a rappresentare. Forse, signor Presidente, sarebbe opportuno un intervento della Presidenza del Senato che facesse proprio questo sentimento di condanna, che mi pare essere stato unanimemente manifestato da tutti i colleghi che si sono espressi finora.

Sono stato direttore del quotidiano «Il Mattino» e ho conosciuto molti aspetti di quel giornale, dei suoi redattori e, ovviamente, anche della città che mi ospitava con molta generosità. Sono stato il primo a recarmi a casa della famiglia Siani e quindi ho una certa dimestichezza con il dovere di un giornale di tutelare e, quando sia possibile, credibile e addirittura doveroso, richiamare l'attenzione delle Forze dell'ordine intorno a dei casi che vanno a colpire la rispettabilità personale ma soprattutto, in questo caso, la responsabilità professionale di un giornalista che si assume il rischio di fare quello che ha fatto la senatrice

vorrei dire che mettere in discussione la legittimità di un provvedimento preso dallo Stato nei confronti di un giornalista che a Napoli - lo ripeto: può significare una cosa grave - questa sì politica e me ne scuso, ma è soltanto un dettaglio - perché scoraggiare, in fondo, la credibilità delle misure che vengono prese nei confronti di quelli che non si adattano a fare giornalismo di giornata, d'accatto, ma si impegnano e rischiano, non solo di perdere la reputazione quando gli si scaglino contro accuse infondate.

Ringrazio tutti i colleghi per i contributi. La Presidenza, anche a titolo personale, esprime la più totale solidarietà, vicinanza e stima

senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. il lavoro svolto dalla Camera dei deputati e poi dalla Commissione giustizia del Senato. Si tratta di una vicenda che definirei per certi versi storica, nel senso che ripetutamente, ogni anno, quando si va verso l'anniversario di gravi e drammatici eventi che hanno insanguinato la vita del nostro Paese, come le stragi della fine degli anni Sessanta, degli anni Settanta e Ottanta e le stragi mafiose degli anni Novanta del secolo scorso,

Se ci limitiamo anche soltanto a ricordare quello che è successo attorno a vicende come la strage di Piazza Fontana o di Piazza della Loggia, la strage di Peteano, la strage di Bologna, attorno al caso Moro e alle stragi mafiose degli anni Novanta del secolo scorso, ci rendiamo conto di come sia quanto mai opportuno e direi necessario, dal punto di vista sociale e politico, prevedere ipotesi e fattispecie di reato specifiche per coloro che in maniera infedele hanno operato contro l'accertamento della verità per queste drammatiche vicende. Da un punto di vista parlamentare, nel corso delle ultime legislature erano stati presentati diversificati disegni di legge che cercavano di mettere ordine in tale materia.

a tutti i senatori, di tutti i Gruppi politici presenti in Commissione giustizia, di avere fattivamente collaborato per creare questo nuovo testo, che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea. Sostanzialmente, proprio per l'esperienza maturata dalle vicende del passato, abbiamo ritenuto di far convergere nel citato disegno di legge le due ipotesi fondamentali, cioè quella di un comportamento materiale delittuoso che viene sussunto sotto la fattispecie della frode processuale secondo determinazioni ed esplicazioni specifiche e quella delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero, davanti al giudice e davanti all'autorità della Corte penale internazionale proprio come attività depistante. A differenza del testo che ci è arrivato dalla Camera dei deputati, che prevedeva una sorta di reato comune generale, in Commissione giustizia del Senato si è ritenuto opportuno configurare il delitto di depistaggio in prima battuta e soprattutto come delitto proprio del pubblico ufficiale, con una pena base, che viene individuata dai tre agli otto anni, e, nei casi particolari di alterazione di documenti e di distruzione di atti sempre al fine di sviare od occultare le indagini,

vengono rese all'interno di procedimenti penali che riguardano i delitti più gravi previsti dal nostro codice penale, e cioè quelli di strage, di terrorismo, di criminalità organizzata e alcuni altri specifici reati indicati. In questo caso, c'è per i pubblici ufficiali la pena dai sei ai dodici anni di reclusione e, per quanto riguarda le dichiarazioni false o reticenti rese, un'aggravante speciale, bilanciata secondo che il comportamento possa configurarsi come dichiarazione falsa, renitente o reticente oppure come favoreggiamento oppure come favoreggiamento nei confronti di colui che ha commesso il reato. Mi limiterei a queste indicazioni sintetiche, vista la richiesta che mi è stata fatta, e magari, durante l'illustrazione dei singoli emendamenti, potrò dire alcune specifiche parole

Signor Presidente, questa proposta è stata abbondantemente elaborata in Commissione della quale fa parte, per il nostro Gruppo, il senatore Di Maggio, che aveva espresso, in linea di massima, un consenso a questo disegno di legge.

si dia vita al consueto processo alle intenzioni, alla fattispecie del reato di opinione. Ho l'impressione - e mi fido, da questo punto di vista, delle valutazioni dei rappresentanti del mio Gruppo che hanno potuto esprimersi in Commissione - che almeno per ora questo testo sia esente da questa preoccupazione. In ogni caso, nel corso della discussione e al momento di valutare gli emendamenti ci sarà migliore e maggiore possibilità di intervenire.

e che affronti una serie di problematiche sulle quali il nostro Paese, negli ultimi trent'anni, si è avvitato in una polemica politica e giornalistica, proprio sul problema della cosiddetta mistificazione della verità o, come indicato in questo provvedimento, il depistaggio. dell'importanza dell'argomento, metto al corrente i colleghi di quanto il capo dello Stato (Napolitano prima e Mattarella dopo) e le alte cariche dello Stato hanno detto negli ultimi due anni, in riferimento proprio a quella che, l'onorevole Bolognesi ha scritto esplicitamente e la senatrice Bonfietti ha ripetuto più volte, sarebbe la materia sulla quale è nata la necessità di introdurre il reato di depistaggio, e cioè

detto: «Sappiamo molto ma non tutto: bisogna insistere, impegnarsi maggiormente per illuminare con la verità gli angoli ancora nascosti di queste vicende, nelle quali si sono intrecciate trame internazionali e nazionali, tradimenti e depistaggi». «Questo è il compito più alto delle istituzioni e delle parti politiche, pretendere chiarezza oltre ogni convenienza». sollecitava «a compiere ogni ulteriore sforzo (...) per giungere ad una esaustiva ricostruzione di quello che avvenne nei cieli di Ustica» e impegnava «tutte le istituzioni a fare la loro parte perché si giunga all'accertamento della verità». E, ancora, Mattarella, l'anno scorso, diceva: «bisogna perseverare nella ricerca tenace di una verità finalmente univoca sull'accaduto» e via così. Appelli solenni delle alte cariche dello Stato per arrivare alla verità. Mi sono impegnato per anni

Naturalmente, mi sono sentito in dovere di informare i colleghi senatori, i deputati e l'opinione pubblica che in quelle carte esplosive ci sono elementi importantissimi per rileggere quegli avvenimenti,

«un raggiro per ingannare la pubblica opinione»; e poi ancora: «Il senatore Giovanardi continua nella sua operazione di disinformazione sulla vicenda di Ustica», «dice il falso»

vedo una certa contraddizione: nei Paesi democratici, dopo trent'anni, si aprono i cassetti e gli storici, i magistrati, l'opinione pubblica e i giornalisti possono accedere; noi, dopo trentasei anni, siamo nelle condizioni di essere accusati di essere dei depistatori di non poter divulgare i contenuti di quelle carte o almeno certi particolari. Certo, chi va a leggere la storia di quel terribile anno 1980 scoprirà, dal libro di Grignetti e dalle dichiarazioni di Zamberletti, che dopo che vennero sequestrati i missili terra‑aria ad Ortona e arrestati un gruppo di palestinesi, insieme a personaggi di Autonomia operaia italiana, si innestò un drammatico cortocircuito

di lasciare circolare liberamente armi sul nostro territorio a condizione che il nostro territorio non fosse colpito da attentati terroristici, come era già accaduto. Il problema fu che quella volta i palestinesi non furono liberati, anzi furono condannati e tenuti in carcere. È, quindi, iniziata una terribile*escalation*, di minacce e rappresaglie, addirittura tese a colpire con precisione vittime innocenti

sulla scia di un certo avvocato Francesco Batticani di Bronte (magistrato? No, avvocato e giudice onorario aggregato), che scrisse, cinque anni prima della sentenza penale, che secondo lui era stato un missile.

e quindi, poiché rimane sul tappeto una sola ipotesi, quella del missile, sulla base del più probabile che non, avendo le parti presentato un solo elemento per spiegare le cose, la Cassazione civile conferma. Però dice che era stato provato il depistaggio. Il depistaggio di chi? Dove è stato provato il depistaggio? Noi stiamo accavallando ed abbiamo accavallato in questi trent'anni tutta una serie di elementi contraddittori, per cui chiaramente e giustamente il capo dello Stato Mattarella dice che bisogna arrivare, su questi fatti, ad una verità univoca e condivisa. Negli Stati civili, quando c'è un incidente aereo - pensate a quello che è capitato sul Sinai qualche mese fa, pensate alle indagini in corso sull'ultimo incidente aereo, pensate a Lockerbie chi è che stabilisce le cause degli incidenti? I periti aeronautici. E una volta stabilita qual è stata la causa che ha provocato la caduta dell'aereo, i magistrati cercano i responsabili. L'Italia invece è l'unico Paese al mondo in cui i periti danno una risposta univoca (è stata una bomba a bordo), ma i magistrati continuano a correre dietro ad ipotesi tipo quella del missile. Ma non solo. Come ho detto, chi sostiene tesi in sintonia con la Cassazione penale e in sintonia con quello che hanno concluso i periti, viene accusato di essere un depistatore e uno che falsifica le carte. Allora io dico: fuori le carte! E chiedo la solidarietà di tutto il Parlamento e del Governo, perché, dopo trentasei anni, si possano conoscere quelle cose che io e alcuni colleghi abbiamo letto.

scritto prima che gli avvenimenti accadessero, compreso il triangolo fra gli estremisti palestinesi, con dietro la Libia e gli autonomi, di cui vengono fatti nomi e cognomi, comprese le città italiane in cui questi

Solo da due anni a questa parte i privilegiati possono leggerle, ma non possono divulgarle. Quindi non possono entrarne a conoscenza gli storici, e i giornalisti: nessuno. Mi sembra allora di vivere una situazione kafkiana. Non dico che ho ragione io e gli altri torto; dico solo che la ragione o il torto si costruiscono attraverso una documentazione che viene messa a disposizione di tutti affinché si possano approfondire tutta una serie di temi che sono veramente significativi per la storia del nostro Paese. C'è chi ha scritto che il lodo Moro non esiste. Se il lodo Moro non esiste, non si capisce perché in pagine e pagine, nelle relazioni su Arafat e i gruppi palestinesi non si faccia altro che parlare di questo accordo,

bisogna arrivare a fare qualcosa di assolutamente condiviso, altrimenti qualcuno sale in cattedra, accusa altri di essere depistatori e qui nasce anche un problema penale. Il depistaggio è una deviazione, una manipolazione dei sospetti emersi in un'indagine: far uscire dalla giusta pista suggerendo tracce fuorvianti; in senso figurato, depistare le indagini. Su alcune cose specifiche sono perfettamente d'accordo con quello che c'è nel testo e, cioè, aggravare le pene per chi commette cose comprensibili; distrugge una prova, falsifica un atto, inquina un ambiente. Tutte cose verificabili.

ente che finalmente in caso di incidente aereo deve andare a vedere tecnicamente come sono avvenute le cose, e gli ho chiesto se era possibile riaprire da parte loro un'indagine, anche tecnica, su Ustica.

non è più elemento di prova. Non si può più fare una perizia su quello che venne recuperato in fondo al mare con spese ingentissime e venne messo a disposizione dei periti, di Taylor, di Lilja, degli svedesi che fecero quella ricerca,

ha permesso di dissequestrare quell'aereo, che era fonte di prova, e lo ha montato male nell'hangar ha depistato? È un depistatore? Lì c'è proprio uno degli elementi fattuali che nella legge sono indicati come depistaggio, alcuni addirittura come frode processuale. Ci sarà una giustificazione e si dirà che sotto pressione di chi lo ha chiesto, il magistrato lo ha concesso: si è fatto però un errore gravissimo perché un fondamentale elemento di prova adesso non lo è più. Al di là degli

che i fatti siano commessi al fine di impedire o sviare un'indagine; ma, colleghi senatori, quando Giovanardi, e non solo lui ma anche gli undici periti internazionali, il processo penale o la Cassazione penale,

hanno sollevato questo problema, chiedendo di andare a vedere le carte, signor rappresentante del Governo, perché il Governo tace? Perché il Governo non ci dice i motivi per i quali, dopo trentasei anni, alcuni di noi possono andare a consultare quelle carte, ma l'opinione pubblica, gli storici e i giornalisti non possono sapere che cosa c'è scritto? Sono io che mi sento danneggiato, perché se dovessi usare il termine «depistaggio», come qualcuno lo ha usato, polemicamente,

Queste sono le ragioni per cui abbiamo presentato degli emendamenti, che illustrerò man mano che verranno richiamati nella discussione dell'articolato.

che però ha una ragione specifica, che sta nella nostra storia. Nella storia del nostro Paese ci sono troppi eventi che costituiscono una ferita, non solo per per il dolore delle persone coinvolte e che sono alla ricerca di una verità che non riescono a trovare; si tratta di una ferita che si allarga e diventa ancora più dolorosa e preoccupante per il concetto stesso di essere partecipi di uno Stato.

Ciò che emerge è un'estrema ramificazione, le difficoltà, la sovrapposizione di testimonianze che vanno in direzione opposta, l'insufficienza dei dati forniti la superficialità nel provvedere prima di tutto ai soccorsi e poi, successivamente, anche nel cercare di perseguire una verità. Ci sono stati 140 morti, le cui rispettive famiglie stanno

In questo modo si sono accreditati e manifestati, pur senza avere il diritto ad un riconoscimento dei fatti e quindi anche delle responsabilità, delle forze, delle ragioni e degli interessi. Nella vicenda Moby Prince si sono mescolati elementi di qualunque natura: dalle navi militari, che in quella notte erano sicuramente ancora nel porto di Livorno,

le famiglie che si recavano in vacanza, il comandante della nave e tutti i portuali. Ne fanno parte anche la comunità di Livorno e tutte le comunità che sono direttamente interessate. In ultima analisi, ne facciamo parte tutti. Il danno che deriva da queste tristi, dolorose e prolungate vicende processuali che non consentono di arrivare alla verità è alla

con un lento rilascio, allontana di fatto i cittadini dalle istituzioni. Il senso del disegno di legge in esame è proprio quello di circoscrivere il reato di depistaggio come

Per questo motivo, nonostante apprezzi moltissimo il lavoro fatto dal relatore in Commissione, che ha consentito una condivisione di molti aspetti del disegno di legge, ho ripresentato un emendamento che,

Non credo che potrò rinunciare a questa modifica perché vorrei sottolineare per tutti che noi dobbiamo affrontare questo problema non solo sotto il profilo dell'istituzione di un reato specifico, ma sotto il profilo culturale, per cui il depistaggio è un'offesa che da chiunque venga fatta, è prima di tutto un'offesa alla potenzialità dello Stato di tutelare tutti i suoi cittadini. C'è anche un altro aspetto che troverete nei miei emendamenti, che può sembrare forte ma che intendo sostenere, ed è l'interdizione dai pubblici uffici. Per me la gravità di questo reato nel caso venga commesso da chi ha un ruolo pubblico, da chi è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, richiede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Noi oggi in questa legislatura e in questo Senato dobbiamo decidere una cosa importante e cioè costruire la personalità di chi si occupa della cosa pubblica, e su questo non ci sono gradazioni.

quale deve essere la qualità di chi si occupa della cosa pubblica a prescindere dall'entità del danno che provoca. C'è un'attitudine, c'è una disponibilità, ed io su questo devo andare a misurare la qualità di chi è incaricato di un pubblico servizio o di chi è pubblico ufficiale. È troppo delicato fare dei distinguo sulla base di una condanna; non è un fatto legato esclusivamente all*'iter* processuale e quindi a quella che sarà la condanna che il giudice deciderà. Questo deve diventare un elemento costitutivo della

se non fossero intervenuti depistaggi, modifiche allo stato dei luoghi e delle cose, distruzione, soppressione, occultamento di oggetti che avrebbero senz'altro aiutato nel difficile percorso di ricostruzione della verità. Una verità che, evidentemente, a qualcuno non sarebbe piaciuta affatto. Esattamente come tante altre volte, forse troppe, abbiamo avuto modo di vedere nel nostro Paese. Dalla strage di Piazza Fontana in poi, omissioni, bugie e distruzione di prove e di documenti hanno impedito

Tra gli atti più eclatanti di depistaggio, non posso non ricordare la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, la cancellazione della memoria del *computer* di Giovanni Falcone, l'introduzione di falsi collaboratori di giustizia nella strage di Via d'Amelio, i depistaggi della strage di Ustica, per non parlare del processo relativo all'accordo tra lo Stato e le associazioni mafiose. Basterebbe questa premessa per considerare favorevolmente l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di depistaggio; potrebbe, infatti, rappresentare un importante strumento per il contrasto alla criminalità, una criminalità non solo di stampo mafioso, ma fatta anche di pezzi deviati delle istituzioni. Il Movimento 5 Stelle è particolarmente vicino a tutte le vittime e a chi da tanti anni lotta per arrivare alla verità che sta dietro alle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese. Per questo motivo siamo favorevoli all'introduzione di questo nuovo reato nel nostro ordinamento, a condizione tuttavia che sia efficace rispetto agli obiettivi che si propone. Quando parliamo di efficacia di una norma, non possiamo non tirare in ballo la prescrizione. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora una riforma dei termini di prescrizione. Ricordo che dall'introduzione della scellerata legge ex Cirielli, la prescrizione ha falciato un milione e mezzo di processi e continua a cancellare procedimenti penali al ritmo di oltre centomila all'anno. Almeno per questo gravissimo reato, il depistaggio, si consideri l'esigenza di non farlo finire in prescrizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A questo scopo abbiamo proposto una modifica all'articolato sulla prescrizione, che ricalca lo stesso regime speciale previsto per i reati di mafia di mafia e ne raddoppia i tempi per tutte le fattispecie considerate nel dispositivo. Si badi bene che se il depistaggio è lo sviamento della pretesa punitiva dello Stato, la prescrizione è addirittura l'estinzione della potestà punitiva dello Stato, cioè è la rinuncia dello Stato a fare giustizia. II testo in discussione potrebbe essere migliorato ulteriormente prevedendo la reintroduzione dell'arresto in flagranza, in caso di falsa testimonianza, con particolare riferimento alla falsa testimonianza del pubblico ufficiale per reati gravissimi. Il falso testimone dovrebbe poter essere perseguito immediatamente, come già avviene nel caso di chi viene sorpreso in flagranza di gravi reati come avviene già, peraltro, in diversi altri Paesi. Il combinato disposto dell'allungamento dei tempi di prescrizione e dell'arresto in flagranza vedrebbe senz'altro rafforzare considerevolmente la portata deterrente della norma. Abbiamo proposto anche di allargare l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a tutte le ipotesi delittuose previste dal provvedimento, estendendola dunque anche ai casi di pene inferiori ai tre anni di reclusione. Se è, infatti, comprensibile e condivisibile la previsione di un grande sconto di pena - dalla metà addirittura fino ai due terzi - nei confronti di chi collabora con l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di depistaggio depistaggio (in considerazione del fatto che questa collaborazione potrà essere utile a scoprire altri reati che stanno dietro al depistaggio medesimo), si considera che l'allargamento della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici possa rappresentare il giusto compromesso

In conclusione, signor Presidente, sono passati sedici anni dalla prima proposta del genere depositata in Parlamento e gli altri tre tentativi che ne sono seguiti sono risultati infruttuosi. Oggi, invece, pare proprio che il Parlamento possa pervenire all'approvazione di questa nuova fattispecie di reato. Chi impedisce, ostacola o svia un'indagine o un processo penale in Italia, con l'introduzione del reato di depistaggio, rischierà una sanzione penale che difficilmente gli consentirà di evitare il carcere.

Questo deriva dall'insegnamento della storia del nostro Paese, avendo rilevato che la grandissima parte dei comportamenti che in questo momento vogliamo divengano delittuosi sono stati posti in essere da coloro che dovevano essere i più fedeli

*(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto raramente in Aula, anche per evitare il rischio della dissipazione delle parole.

della strage di piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Una vicenda che, come documentato in sede giudiziaria, certamente annovera attività di depistaggio. Non c'è dubbio che una distinzione vada posta tra la necessità di perseguire il depistaggio, inteso come fatto concreto e materiale,

anche io, come alcuni colleghi, ho potuto consultare, grazie al fatto di essere membro della "Commissione Moro", i documenti cui il collega Giovanardi fa riferimento.

Mi pare che una obiezione di fondo sia possibile rivolgere al collega Giovanardi, e gliela propongo senza alcun pregiudizio o preconcetto.

Innanzitutto, in quelle carte certamente si fa riferimento a un quadro politico dentro il quale è possibile riconoscere una politica da immunità pattuita. Rimandare esplicitamente ad un lodo Moro che, fino a prova contraria, sulla base di riscontri documentali, oggi non è ancora stato individuato, a me pare perlomeno imprudente. È possibile, certamente, lo ribadisco, parlare di una politica da immunità pattuita e questo emerge dai documenti. Per il momento, però, allo stato delle conoscenze attuali, non mi pare sia possibile spingerci oltre.

che quelle carte sono significative e rilevanti sotto il profilo dell'interpretazione storica di una particolare stagione e di uno specifico momento dello sviluppo della politica italiana.

In realtà due sono le obiezioni che si possono sollevare alle conclusioni che il collega, secondo me in modo eccessivamente precipitoso, trae.

Il collega Giovanardi solleva un problema vero, che è quello della desecretazione. Al di là dei meriti che indubbiamente il presidente Renzi ha acquisito sotto il profilo della desecretazione degli archivi,

condizioni del clima politico, non sia opportuno rendere conoscibili queste carte. Posta così la questione, credo che l'interrogativo sollevato dal collega Giovanardi sia legittimo e condivisibile.

degli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103, altrimenti esprimo parere contrario. La questione fa riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna, per quanto riguarda il testo proposto, dovrebbe essere superiore ai tre anni. Si esprime il predetto parere perché, pur condividendo le sollecitazioni e lo spirito di questi emendamenti, rilevo che ci sono profili di illegittimità costituzionale, in quanto esiste tutta una serie di reati molto più gravi per i quali non si pone questo tema, quindi il trattamento diversificato creerebbe profili di illegittimità costituzionale.

parimenti c'è un invito al ritiro o l'espressione di un parere contrario, in quanto si tratta di un tema che verrà affrontato proprio in questi giorni dalla Commissione giustizia e perché si inserisce

profili di ragionevolezza e di corrispondenza d'ordine costituzionale, non possono essere inserite per evitare trattamenti di disuguaglianza. Invito quindi al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Non essendo stato stabilito un orario di chiusura della seduta, ma essendo la Presidenza orientata - se supportata dall'Assemblea - a chiudere la seduta dopo la conclusione di questo provvedimento, prima facciamo, meglio è.

su «National Geographic» con le dichiarazioni in inglese di Taylor, che in pratica conclude dicendo: «Noi abbiamo scoperto la verità, ma i magistrati non se la vogliono sentir dire». che quattro anni di lavoro degli undici più grandi periti internazionali secondo lui erano contraddittori. Il dottor Priore venne sconfessato totalmente nei tre gradi di giudizio. quindi, è un po' più complessa: qual è la verità? È quella di un magistrato che non sa nulla di tecnica o degli 11 più grandi periti del mondo? Chi è il depistatore? Queste Queste vicende, se vanno nel senso indicato dalla collega, possono penalizzare e incriminare chiunque sostenga una tesi diversa. Caro senatore Corsini, so anch'io

intervengo sull'ordine dei lavori. Visto l'atteggiamento collaborativo del collega Giovanardi, chiedo se può cortesemente estrarre la tessera del suo vicino di banco, senatore Formigoni, assente.

poiché stiamo parlando di depistaggio e di segreti, è evidente che non troveremo mai un documento scritto e firmato da Aldo Moro sulla questione

Signor Presidente, dico sin d'ora che il Gruppo della Lega Nord è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che introduce nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio. prevede la reclusione per il pubblico ufficiale che, al fine di impedire o ostacolare un'indagine o un processo penale, inquini le prove, fornisca informazioni false e depisti in definitiva le indagini. È evidente quindi che si dà risposta, con questo provvedimento, alle richieste di molte di molte associazioni di vittime di reati molto gravi, come le stragi terroristiche, che chiedevano da tempo l'introduzione di questo reato. Noi riteniamo che questo provvedimento darà nuovi strumenti agli inquirenti e alla magistratura non solo per colpire i reati, ma soprattutto per togliere il velo di omertà rispetto a tanti segreti e a tante non verità che hanno caratterizzato eventi tragici che hanno colpito il nostro Paese. È una scelta giusta, soprattutto per rispetto delle vittime di questi avvenimenti e per rispetto delle loro famiglie. Ci auguriamo naturalmente che tale provvedimento abbia un'efficacia reale e che non rappresenti una scelta di comodo, solo per evidenziare l'attenzione della politica rispetto alle richieste di giustizia delle associazioni delle vittime delle stragi, private ancora oggi del diritto alla verità. Dobbiamo però rimarcare un atteggiamento molto contraddittorio da parte di questa maggioranza e di questo Governo. In questi ultimi tre anni, infatti, sono stati introdotti nuovi reati, reati, che vogliono dare risposte ad alcune associazioni. Mi riferisco ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, trasporto e abbandono di rifiuti radioattivi, impedimento ai controlli e omessa bonifica. nuovi reati introdotti da questa maggioranza e da questo Governo; e così anche è stato introdotto il reato di omicidio stradale, per dare risposta alle associazioni delle vittime. Oggi c'è un nuovo reato, che riguarda il depistaggio, per dare risposta alle associazioni delle vittime delle stragi. Ebbene, noi riteniamo contraddittorio il fatto che questo Governo introduca continuamente nuovi reati, promuovendo evidentemente la possibilità di celebrare nuovi processi, e dall'altra abbia varato, in tre anni, cinque provvedimenti svuota carceri. Quindi da una parte aggrava ancor di più i tribunali di nuovi procedimenti e dà risposte di immagine alle associazioni di vittime della giustizia, ma nel concreto questo Governo e questa maggioranza hanno messo in libertà migliaia di delinquenti, migliaia di delinquenti, che erano stati messi in carcere dopo lunghe indagini e dopo essere stati oggetto di processi. Quindi si dà la possibilità a rapinatori, spacciatori e truffatori di agire liberamente sul nostro territorio, perché l'unica risposta rispetto al problema del sovraffollamento delle carceri è stata quella di svuotarle, mettendo in giro delinquenti che circolano liberamente sul nostro territorio, rendendo il nostro Paese la sede ideale di bande organizzate e dedite ai furti nelle abitazioni.

un Parlamento, una maggioranza e un Governo che dicono «no» alla legge per riformare la legittima difesa, per evitare che chi è vittima dei delinquenti non lo diventi anche della giustizia italiana. che non siamo assolutamente in linea con l'azione del Governo sulla giustizia, ma rispetto a questo particolare provvedimento assicuriamo il nostro voto favorevole.

l'importanza dell'argomento. Prendo atto del fatto che, salvo il collega Corsini, in maniera elegante, nessuno dei colleghi si è associato alla mia richiesta al Governo perché dopo trentasei anni questi documenti vengano resi pubblici. Dopodiché, il 27 giugno sentiremo il Capo dello Stato fare il solito solenne appello alla ricerca della verità e all'impegno delle istituzioni per la verità. Sentiremo i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato dire che faremo di tutto, ma prendo atto che in questa Assemblea nessuno dei senatori si è posto il problema, dopo trentasei anni, mentre si discute di depistaggio, di andare a vedere le fonti per capire eventualmente chi e che cosa depistava. Allo stato degli atti il vero depistatore mi sembra il Governo, che si rifiuta di rendere pubblici atti decisivi per la ricostruzione dell'argomento di cui abbiamo parlato stamattina.

di colpire con pene gravissime i supposti depistatori, mentre il Senato si rifiuta di associarsi alla mia richiesta, affinché il Governo dopo trentasei anni renda pubbliche delle carte, che possono essere interpretate in maniera diversa, caro Presidente - dal ma bisogna che vengano rese pubbliche. Altrimenti come facciamo a confrontarci rispetto a tutte le ipotesi di fantascienza, con i registi che si sono arricchiti coi film,

ci sono i fischi della piazza, perché è uno scandalo che non si vengano a sapere le cose coperte e, oggi che abbiamo la dimostrazione che le cose continuano ad essere coperte e non sono divulgabili, nessuno dice niente? A me sembra di sognare.

di come questi abbiano avuto a che fare anche con elementi di difficoltà della democrazia di questo Paese. Credo che la domanda che ci poniamo, cioè perché solo oggi viene messo in luce questo provvedimento, la dica lunga su quale sia stato il clima in questo Paese in tutti questi anni, da Portella della Ginestra in poi, passando per la strage di Stato di Piazza Fontana, fino alle stragi di Brescia, Bologna e a tutto quello che è accaduto negli anni passati. Ebbene, l'introduzione del reato di depistaggio ci sembra davvero il minimo sindacale, se posso dire così. Voteremo ma pensiamo che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo. sembra esprimersi sostanzialmente all'unanimità in occasione dell'approvazione di un disegno di legge. Anche in questa occasione, sono ben lieto di annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge che introduce finalmente il reato di depistaggio nel nostro ordinamento penale. Rimane solo qualche perplessità in relazione ad un paio di emendamenti che il Movimento 5 Stelle aveva proposto proposto anche in Assemblea. Ho ascoltato la replica del relatore, ma francamente tutti i dubbi non sono stati sgombrati. Mi riferisco precisamente alla circostanza che noi

delle osservazioni certamente legittime, ma occorrerebbe ricordare che vi sono altri casi, già previsti dal nostro codice penale, in cui, al di là dell'entità della pena (nel caso del disegno di legge si prevede che l'interdizione scatti solo con una condanna superiore a tre anni di reclusione), la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici scatta a prescindere dalla quantità di pena erogata. Mi riferisco a quanto già disposto nell'articolo 317 317 del codice penale, che prevede per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla pena erogata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici:

dalla nuova norma e del bene giuridico che qui il legislatore vuole tutelare, che è quello di una verità processuale che possa essere inquinata e attentata il meno possibile soprattutto da parte dei pubblici ufficiali che

perpetua sarebbe meritevole di accoglimento da parte di questo ramo del Parlamento. Vedremo se alla Camera si vorrà avere un ripensamento perché, lo ripeto, non sarebbe una novità assoluta e quindi a livello di sostenibilità costituzionale continuiamo a pensare che sarebbe stato possibile appoggiarla. Anche la proposta fatta in Aula, attraverso un altro emendamento, relativa alla proposta di raddoppiare i termini prescrizionali per il reato di depistaggio è stata bocciata perché il relatore ci ha fatto presente che effettivamente all'esame della Commissione giustizia vi è la riforma del procedimento penale che prevede delle formule variegate di allungamento della prescrizione. Tuttavia, credo che se avessimo approvato la norma che avrebbe disposto il raddoppio dei termini prescrizionali per il reato di depistaggio, anche in sede di coordinamento in futuro si sarebbe potuto sciogliere ogni eventuale discrasia normativa.

non è condizionata dal Governo si riescono ad individuare delle soluzioni tecniche che consentano di arrivare all'unanimità.

Abbiamo individuato insieme un reato proprio. Non voglio qui ripetermi e vorrei soltanto soffermarmi su alcuni aspetti emersi nel dibattito e che lasciano ancora dei dubbi in qualcuno. Questa

una responsabilità penale di maggior gravità rispetto a quella applicata fino ad oggi per avere una maggiore deterrenza di devianze.

che bisogna fare un'ulteriore indagine. Su questo non c'è dubbio. Io posso intervenire sui giornali o con un libro e sostenere che una determinata indagine o che la sentenza del tribunale o della corte d'appello è sbagliata.

dichiari una cosa diversa dal vero oppure si faccia falsa testimonianza in giudizio. Avendo pure conoscenza, poiché faccio parte della "Commissione Moro", di atti segreti,

nonostante siano stati fatti accertamenti giudiziari e condanne. Ciò non significa che non potrò esprimermi; non è assolutamente vero!

per questo vuoi condannarli? Non esiste! Questa legge mira ad altro. Facciamo in modo che i pubblici funzionari non intervengano nella fase delle indagini non cerchino di sviare l'attenzione del pubblico ministero dalla ricerca di determinati filoni di indagine, giusti o sbagliati che siano. Una cosa è la critica ed un'altra è l'intervento per deviare. Noi abbiamo avuto episodi di devianza, ma non dobbiamo confondere.

Quegli atti devianti oggi diventano depistaggio, ma non si modifica alcunché rispetto all'attuale situazione. L'unica vera modifica riguarda la maggiore gravità e la maggiore individuazione dei comportamenti concreti che possono determinare il reato di depistaggio e, quindi, determinare, di conseguenza, una deterrenza e una astensione dei pubblici ufficiali da comportamenti del genere. Per questa ragione voteremo a favore Presidente, il Partito Democratico voterà convintamente questo disegno di legge che finalmente inserisce la condotta penalmente rilevante di depistaggio nel nostro codice. Devo ringraziare l'onorevole Bolognesi alla Camera e il senatore Lo Giudice qui al Senato che, anche in questa legislatura, presentando dei disegni di legge con diverse firme, sia di deputati che di senatori, hanno spinto perché si arrivasse a questo importantissimo risultato. Cari colleghi, la storia del nostro Paese è chiara. Le stragi si sono consumate. Ricordo ai colleghi piazza Fontana, piazza della Loggia, Peteano, Bologna, Ustica,

qui non ci stiamo occupando delle opinioni che ognuno di noi ha intorno a queste stragi. Non ci stiamo occupando delle ricostruzioni giornalistiche o storiche delle stragi. Esistono delle Commissioni d'inchiesta che hanno lavorato, e alcuni lavori sono tuttora in corso, come nel caso della "Commissione Moro". Cari colleghi, qui ci stiamo occupando semplicemente delle condotte penalmente rilevanti che ostacolano, impediscono e deviano il corso della giustizia, dalle indagini al dibattimento a tutte le fasi processuali. Di questo ci stiamo occupando, perché una democrazia deve poter avere al suo interno delle dinamiche politiche anche roventi e conflittuali in alcuni momenti storici. Mai però si deve utilizzare lo strumento delle stragi per provare a condizionare e deviare il corso della democrazia. Cari colleghi, anche per le dinamiche sociali, in alcuni momenti vi sono dei conflitti fortissimi su questo livello importante di democrazia. Anche in questo caso, però, mai le stragi devono diventare uno strumento

una fattispecie penalmente rilevante. Colpiamo i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, perché all'interno dello Stato mai un servitore dello Stato deve imboccare una strada che possa impedire la ricostruzione penalmente rilevante dell'accertamento della verità. Naturalmente, colpiamo anche i cittadini comuni, prevedendo delle circostanze aggravanti che partecipano a questo odioso reato. Ecco perché, cari colleghi, possiamo votare convintamente a favore di anche una larga convergenza, finalmente il nostro Paese al Senato ha trovato la via giusta. Ci auguriamo che la Camera

ha precorso i tempi. Purtroppo è mancato; comunque, prima che la malattia avesse ragione del suo fisico molto forte per la seconda volta

in occasione della prima ondata di immigrati nel biellese ha predisposto l'accoglienza e l'ospitalità per gli immigrati, ha fondato delle cooperative sociali nei quartieri popolari. Aveva iniziato da lì c'era il seme per far lavorare i disabili all'interno delle cooperative e per includerli nella vita della comunità. Poi ha creato una casa famiglia nella parrocchia, dove è stata accolta una bimba *down*,

ci sono state delle conquiste; nel 2003 ha costituito il "dopo di noi" per lanciare un cammino di promozione sociale delle persone con disabilità nei contesti di normalità. Leggo solo la lettera che è stata inviata a Pasqua, molto prima

Dio ha messo delle cose meravigliose che noi dobbiamo imparare a vedere e far emergere». A tanti papà (perché lui è stato papà di Loredana per tanto tempo) e a tutti i genitori, ai tanti don Egidio che hanno voluto fortemente che ci fosse il "dopo di noi" ma anche il "durante noi", io dedico

finestra") del 2013, che riguarda la situazione del tratto ferroviario Terracina-Priverno Fossanova, ormai chiuso dal 12 settembre 2012. 2012. Qualcuno potrebbe chiedersi perché sollecitare una interrogazione di quasi tre anni fa, ma la spiegazione è molto semplice. Nella giornata di ieri il ministro Delrio, intervenendo durante un evento tenutosi in un hotel di Terracina, a sostegno del candidato sindaco del Partito Democratico - ma questa chiaramente è una casualità ha sostanzialmente confermato stanziamenti milionari che dovrebbero servire alla soluzione, tra le altre, anche di quella annosa e deprecabile situazione, da me segnalata al Governo già nel luglio del 2013. Lo stesso orientamento hanno le dichiarazioni fatte nella stessa sede dall'assessore alle infrastrutture della Regione Lazio Refrigeri: «Abbiamo un treno che si ferma per mancanza di sicurezza? No a inutili promesse. Abbiamo cercato di capire, consultato l'unità di crisi di palazzo Chigi, abbiamo fatto un progetto con RFI, e deciso: quella tratta va percorsa, è utile e sostenibile». E ancora: «La politica parla con gli atti» e dunque «rimane in silenzio fino a quando non può dare garanzie». io sono estremamente lieto di apprendere queste informazioni grazie a un evento di partito. Ma sarebbe necessario e corretto, per allontanare i dubbi dei malpensanti che potrebbero invocare la classica boutade preelettorale, che il tutto venisse formalizzato anche in una sede più opportuna, magari in quest'Assemblea parlamentare. Rinnovo quindi la richiesta che il Governo venga a rispondere alla mia interrogazione ufficializzando le proprie intenzioni, perché altrimenti, parafrasando le parole dell'assessore Refrigeri, potremmo dire che la politica rimane in silenzio fino a quando non inizia la campagna elettorale.

nei giorni passati, sulla a dir poco scellerata e sciagurata idea di chiudere il presidio ospedaliero dell'isola di Procida. è salita alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni non per le sue, peraltro, ben conosciute bellezze, ma per il fatto che è stata giustamente attraversata da molte manifestazioni di protesta della popolazione procidana, sdegnata, per l'appunto, e del tutto giustamente, in maniera finanche sacrosanta, per la davvero sciagurata idea, contenuta nel piano ospedaliero, di ridimensionare fortemente il presidio ospedaliero, riducendo il numero dei posti letto da nove a tre, immaginando soltanto un minimo primo soccorso e non più la diagnostica. Procida è un'isola e, quindi, è scollegata dalla terraferma. Bisogna attraversare il mare, ovviamente, quando una persona non sta bene, e capite bene tutti come sia davvero insensato e incredibile, in una situazione come questa, non solo non fare quello che andava fatto, e cioè potenziare il presidio ospedaliero, ma all'opposto, depotenziarlo. C'è stata qualche davvero minima, purtroppo, apertura nel corso delle ultime ore, anche a seguito di una giusta e sacrosanta mobilitazione che, peraltro, oltre ai procidani ha attraversato anche il *web*, con decine di migliaia di messaggi di solidarietà. Vorrei dire in quest'Aula che detta vicenda va

dell'isola, di lasciare il presidio ospedaliero così com'è; anzi, se possibile, di migliorarlo. Parliamo infatti di un'isola che ha 10.000 abitanti, che già non sono pochi, durante l'anno, e che arriva ad averne

ci sembra una scelta completamente insensata. Quindi, chi l'ha fatta deve cambiare rapidamente idea, perché offende non soltanto i cittadini di Procida ma tutte le persone di buonsenso di questo Paese. Signor Presidente, il calcio per gli italiani - e forse non solo per loro - è lo sport più bello del mondo, per i giovani di certo, per i quali è il mondo del successo e dell'affermazione, ma anche il contesto in cui spesso vengono proiettate speranze e ansie e talvolta anche rabbia, frustrazione e disperazione. Lo si voglia o no, il calcio e la giustizia sportiva assumono talvolta una rilevanza che travalica i confini della cronaca sportiva e finiscono per diventare occasione di contestazioni e scontri tra tifoserie, che spesso vedono coinvolte anche le Forze dell'ordine. Per questo è importante oserei dire fondamentale - che i verdetti sul campo siano conseguenze solo di una supremazia o di una maggiore fortuna di una squadra sull'altra e soprattutto che, al netto degli errori umani, sempre possibili, sia garantito il principio di imparzialità dell'arbitraggio, perché ciò è condizione indispensabile e garanzia necessaria di legalità e correttezza. Così non è stato - mi viene da dire ancora una volta - per la squadra del Livorno Calcio, impegnata nell'ultima partita di campionato nella serie cadetta, nella sfida diretta con il Lanciano per l'accesso ai *play out* con la Salernitana di Lotito ed evitare la retrocessione diretta. È accaduto che, per un fallo platealmente inesistente del portiere del Livorno, sia stato concesso un rigore ed espulso il portiere stesso. Mancavano meno di quindici minuti alla fine e il Livorno vinceva agevolmente per due a zero. Il risultato è stato così ribaltato in pochi minuti. il caso vuole che la giustizia sportiva, prendendo atto del comportamento scorretto del giocatore, abbia giustamente comminato due giornate di squalifica, per simulazione di fallo, al giocatore del Lanciano che aveva ottenuto quel rigore determinante per l'esito della partita. Ritengo che anche l'arbitraggio e il verdetto debbano in maniera corrispondente prenderne atto. Segnalo, per altro, che il Lanciano Calcio era stato già sanzionato per gravi irregolarità amministrative con la perdita di cinque punti, poi inspiegabilmente ridotti a due in appello. Per la delicatezza delle implicazioni che la vicenda può suscitare e nel raccomandare la massima attenzione a tutti i soggetti coinvolti, ho depositato oggi stesso - e ne informo con questa comunicazione la Presidenza e l'Aula un'interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio in qualità di Ministro allo sport, sollecitandone una pronta risposta e auspicandone un conseguente intervento.